come già comunicato ai Gruppi per le vie brevi, nella seduta di domani, alle ore 15,30, la Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, onorevole Stefania Craxi, renderà un'informativa sulla situazione in Siria. I Gruppi potranno intervenire per cinque minuti ciascuno.

che «non può essere effettuata se non in presenza di ragionevoli dubbi in ordine alla persistenza delle condizioni medesime»;

superfluo perché, quando si prevede che la verifica della sussistenza «non può essere effettuata se non in presenza di ragionevoli dubbi», vuol dire che si tratta

le parole: «minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica» (articolo 20

È vero che nella direttiva 2004/38/CE si parla di interesse fondamentale della società, però è un concetto giuridico che non si sposa con il nostro ordinamento in quanto noi abbiamo dei diritti fondamentali e non degli interessi fondamentali. Inoltre, il collegamento alla società intesa in senso generale non va bene. norma di cui al decreto è quella corretta: «minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica». Questo interesse fondamentale noi lo abbiamo trasformato in questi due concetti, che sono concetti calzanti. Anche sull'emendamento 1.2 1.2 formulo un invito al ritiro oppure un parere contrario.

perché si riallaccia ad una norma nella quale è stato sostituito il potere del Ministero dell'interno, per determinati allontanamenti, con il potere del prefetto. Ora questo appare più logico, perché affidare i provvedimenti di allontanamento per motivi di ordine pubblico al Ministero dell'interno è in un certo senso ridondante.

territorialmente competente quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato.

Come si riallaccia l'emendamento 1.3? Si riallaccia perché si vorrebbe ripristinare l'ordine pubblico nella

al comma 1

Presidente, mi sembra evidente l'atteggiamento del relatore di auto-ostruzionismo, che dovrebbe cessare subito, perché non è degno della funzione che è chiamato a svolgere. *(Applausi dal

L'emendamento 1.3 è molto complesso, anche se è di una sola riga! Allora, per arrivare ad una conclusione, volevo spiegare che avevo ben capito cosa era stato scritto.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, annunciando il nostro voto contrario a questi emendamenti, vorremmo anche spiegare le motivazioni di un tale voto. Stiamo Stiamo intervenendo, con l'articolo 1 di questo decreto-legge, su una materia estremamente delicata, qual è quella relativa alla libera circolazione dei cittadini comunitari, ed interveniamo modificando il decreto‑legislativo del 6 febbraio 2007, n. 30. Come sapete, è un provvedimento che è stato modificato all'inizio di questa legislatura, inserito alcune norme particolarmente importanti che hanno avuto effetti positivi in termini di allontanamento di cittadini comunitari che hanno commesso gravi reati e che, quindi, rientrano nelle tipologie e nelle categorie espressamente indicate I senatori dell'opposizione propongono un affievolimento degli strumenti di allontanamento coattivo dei cittadini comunitari che non possono però trovarci concordi. Abbiamo sempre assunto una posizione molto chiara, sin dall'inizio di questa legislatura; ovviamente, non contestiamo il diritto alla libera circolazione dei cittadini comunitari, anche di cittadini comunitari che fanno parte di Paesi che sono entrati da poco nell'Unione europea, ma abbiamo una posizione di estremo rigore,

Voi sapete che il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, è un provvedimento che dà attuazione alla direttiva

non diventino un onere eccessivo per il sistema sociale dei Paesi che li ospitano. Questo è un punto che, formulato in questi termini, può presentare delle criticità, ma indubbiamente per noi diventa un caposaldo a cui attenerci anche ai fini del relativo allontanamento, e il provvedimento interviene anche su questa materia. Certamente un punto essenziale della direttiva e del decreto legislativo è quello relativo ai motivi di sicurezza pubblica che stanno alla base dei provvedimenti di allontanamento. Alla luce di queste motivazioni e della necessità di tener fermo l'indirizzo che abbiamo adottato sin dall'inizio di questa legislatura, annuncio il nostro voto contrario agli emendamenti presentati dall'opposizione.

previsione contenuta nel testo che stiamo esaminando. Tra l'altro, la formula proposta lascia parecchi dubbi, perché resta nel vago e non consente la la possibilità di fare delle verifiche vere e proprie. Oltretutto, in questi casi non ci troviamo a che fare con situazioni di ordinaria burocrazia, ma con situazioni difficili, a volte di emergenza, e non credo sia positivo stabilire norme rigide

quanto proposto va considerato nel contesto del provvedimento e, alla luce di questo contesto, occorre considerare anche che il relatore ed il Governo hanno dato parere contrario.

se siamo sinceri, siamo costretti ad ammettere che potrebbe essere la descrizione perfetta del danno subito dai 25 immigrati stivati dentro la sala macchina, gasati dalle emanazioni tossiche e tenuti dentro dagli aguzzini che li hanno rinchiusi. Questo sia detto di passaggio. Il senso dell'emendamento è che l'espressione "incolumità pubblica" è attinente ad una visione delle cose come potrebbe essere quella, sia pure rispettabilissima, di un questore che affronta le ragioni dell'incolumità pubblica; dal nostro punto di vista, è di gran lunga preferibile il testo della direttiva: «una minaccia reale ed attuale,

che ne sia dichiarata l'espulsione, di avvalersi del diritto di richiedere asilo o protezione umanitaria. La differenza, come il Governo sa, è molto rilevante perché il fatto di aver potuto presentare immediatamente la richiesta di protezione umanitaria, come è diritto di ciascuna persona se pensa di poterlo fare, dà diritto a queste persone di non essere rinchiuse in un centro di identificazione e di espulsione in condizioni di privazione di libertà, ma di essere accolte in un centro di accoglienza, che è una situazione totalmente diversa. diversa. Inoltre, con l'emendamento si chiede che, prima di adottare un provvedimento di espulsione, allo straniero sia comunque illustrata la possibilità di essere ammesso a programmi di rimpatrio assistito. Il senso di questa proposta mi pare evidente.

possa rappresentare in alcun modo un costo: si può essere a favore o contro l'emendamento, ma non mi pare che esistano questioni di costi o di copertura che lo possano riguardare. Per questo, anche se

Peraltro, il testo del decreto-legge che il Governo ci propone è in netta contraddizione rispetto ai contenuti, chiari e precis,i della direttiva comunitaria. È per questo che noi, come Partito Democratico, abbiamo presentato una serie di emendamenti al testo dell'articolo 3 del decreto-legge, da un lato proponendo, con l'emendamento 3.100 della senatrice Marinaro, un testo alternativo e realmente attuativo della normativa comunitaria, dall'altro prospettando singoli e specifici emendamenti volti a migliorare comunque il testo del decreto-legge. Illustrerò ora sinteticamente i criteri che ci hanno spinto all'elaborazione di questi emendamenti migliorativi. evidente la contraddittorietà della politica del Governo in questa materia con quanto sostenuto da questa stessa maggioranza politica in ambito europeo. In primo luogo, ricordo che la specifica direttiva rimpatri era stata presentata a livello comunitario dall'allora commissario europeo Franco Frattini, attuale Ministro degli affari In secondo luogo, ricordo che questa direttiva era stata fortemente voluta dal Gruppo del PPE, di cui il PdL fa parte nel Parlamento europeo. Infine, non pare inutile rammentare che questa direttiva è stata sostenuta, approvata e votata dal ministro Maroni nel Consiglio dei ministri dell'interno dell'Unione europea. Poi cosa è successo? Per quale motivo il Governo italiano da allora si è rifiutato di recepire e di dare applicazione a quella direttiva, facendo per di più scadere il termine del 24 dicembre 2010 e creando così le premesse sia per un'ennesima procedura d'infrazione, già avviata dalla Commissione europea, sia per una condanna da parte della Corte di giustizia evidente che l'emanazione di quella direttiva del 2008 ha sancito il fallimento istituzionale dell'approccio repressivo di questo Governo sulla questione dell'immigrazione, soprattutto rispetto allo spirito e alla *ratio*, assolutamente agli antipodi rispetto alle direttive e ai principi europei. È per questo che le norme di cui all'articolo 3 di questo decreto-legge si avviluppano al loro interno nel tentativo di limitare il più possibile l'impatto della direttiva, di recepirne soltanto alcune parti, ma soprattutto di invertirne la logica politica e sociale. È questo uno dei motivi per cui riteniamo che il decreto-legge in esame non risolverà il già vasto contenzioso in materia con l'Unione europea. Ma quello che più ci preoccupa, oltre a disposizioni correttive e integrative di non facile lettura, è la carenza di un disegno organico e di norme in grado di governare veramente e seriamente il fenomeno migratorio, così come la mancanza di rispetto dei diritti fondamentali della persona, di tutte le persone. In questo il vostro decreto-legge si allontana dalla civiltà europea perché si concentra per davvero solamente sulla coazione, sulla forza, sulle espulsioni coatte, mentre considera partenze volontarie e rimpatri - di cui parliamo nei nostri emendamenti - delle mere eccezioni, dimenticando che la Corte di giustizia dell'Unione europea ancora nell'aprile di quest'anno ha ribadito la necessità di prevedere la successione graduale delle fasi della procedura di rimpatrio, dalla misura minima e meno restrittiva della libertà personale fino alla misura più restrittiva, come *extrema ratio*, ma con limitazioni ben precise, comprese quelle temporali. In ciò con il vostro decreto-legge viene stravolta la logica politica e sociale, vengono violate le norme fondamentali, anche costituzionali, e vengono disattesi i principi e gli obiettivi europei. I nove emendamenti che ho citato fanno riferimento a questo contesto europeo e pertanto ne chiediamo l'approvazione.

Noi riteniamo che alcuni di questi emendamenti abbiano pregio, ma, o sono troppo complessi (per esempio, ce ne sono un paio della senatrice Marinaro e di altri senatori che riformano

l'accoglimento di alcuni dispositivi di ordini del giorno modificati; stamattina, mi pare, sono stati tutti accolti, salvo quello sul quale è stato chiesto il voto dal collega Pedica. Quindi, come già si era discusso a lungo in Commissione, noi certamente siamo favore - lo abbiamo già fatto - le proposte dirette a consentire l'accesso dei giornalisti nei centri di identificazione a verificare l'applicazione delle nuove norme al fine di pervenire a una riduzione del termine massimo di trattenimento. Ci sono degli ordini del giorno che parlano espressamente di un monitoraggio per verificare

attraverso una serie di passaggi, arriva espressamente ai diciotto mesi; siamo i primi a sperare che attraverso un monitoraggio si possa far scendere questo termine e arrivare a un numero di mesi non così elevato. non dimentichiamo mai che chi viene trattenuto in un centro di identificazione è colui che non vuole in alcun modo dimostrare documentalmente la sua identità o dire il proprio nome. Questo non voglio considerarlo un comportamento non

perché noi tutto possiamo fare, prevedere ogni tipo di provvidenza utile, tentare di integrare, di tenere, di dare permessi normali o di carattere umanitario, ma non ci possiamo permettere di avere sul territorio persone non identificate, perché queste ultime possono diventare

dai Gruppi* *PdL e PD).* Se però il senatore Legnini è riuscito a impedirmi di sviluppare il mio ragionamento su un emendamento, credo che un atteggiamento di questo genere non sarebbe gradito.

esprimo parere contrario sulle premesse. Per quanto riguarda il dispositivo, chiedo di eliminare dal testo le parole «e nel primo provvedimento utile».

tutte le modifiche, anche legislative, necessarie a recepire nell'ordinamento italiano lo spirito e la *ratio* della direttiva al fine di rendere più accessibile la partenza volontaria nell'ambito della disciplina di rimpatrio dei cittadini dei Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare».

«predisporre tutte le misure necessarie affinché la disciplina dell'allontanamento e del trattenimento sia caratterizzata dalla medesima gradualità delle misure adottabili a partire da quelle prioritariamente indicate dalla direttiva, quali la partenza volontaria, fino a giungere alle misure più coercitive, al pari di quanto disposto dall'intero articolato della direttiva». Sull'ordine del giorno G3.106, esprimo parere favorevole, comprese le premesse.

un emendamento dell'opposizione che ha ulteriormente consentito di chiarire che non può essere comunque superato il termine massimo dei 18 mesi.

Onorevoli colleghi, è pervenuta alla Presidenza una richiesta, a prima firma del senatore D'Alia, per la votazione a scrutinio segreto degli emendamenti 3.3, 3.22, 3.36, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43 e 3.44. Alla luce della costante prassi applicativa dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la Presidenza ritiene ammissibile tale richiesta, che andrà nuovamente supportata al momento della votazione dei singoli emendamenti. Stante

aggravare la situazione e, quindi, ingolfare i CIE, già gravati per una serie di ragioni di cui si è già parlato. Misura grave per la libertà personale e, anche dal punto di vista operativo, misura inefficace e inefficiente, visto che si potrebbe provvedere

sostituire il primo ed il secondo periodo con il seguente: valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima allo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni».

dà una *chance* in più agli stranieri in condizione di andarsene volontariamente a casa propria.

Vorrei poi fare una brevissima premessa dicendo: meno male che c'è l'Europa, così questo Governo deve, sia pure *obtorto collo*, adeguarsi alla direttiva europea. Certo, il ministro Maroni soffre un po':

per la stragrande maggioranza da Paesi governati dalla destra e dal centrodestra. Questo vuol dire forse che tali Paesi hanno un senso civico, e un senso di civiltà, per quanto riguarda le migrazioni, un po' più elevato del nostro. L'emendamento 3.22 riguarda l'irregolare al quale sia stato concesso un termine per la partenza volontaria. L'emendamento sopprime seguente dizione: «il questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilità dell'assegno sociale Ebbene, si considerino tre aspetti. Come fa un irregolare, che ha un lavoro irregolare a nero, ad avere denaro di fonte lecita, quando probabilmente il suo datore di lavoro, che gli ha dato lavoro a nero,

Se il rimpatriando rimpatria subito, perché chiedergli fino a tre mensilità dell'assegno sociale? C'è evidentemente una sproporzione tra la durata del tempo che gli viene assegnata prima di partire e la richiesta economica che gli viene avanzata. avanzata. L'ultimo aspetto riguarda il fatto che chi non ha risorse forse è anche colui che ha più voglia di rientrare nel proprio Paese e meno *chance* di rimanere nel Paese nel quale si si trova irregolarmente. Quindi, l'emendamento in esame cancella questa contraddittoria e inutile disposizione. Infine, ne cancella anche un'altra, perché

penali la violazione delle prescrizioni da parte dello straniero, nelle more dell'espulsione, prevedendo la competenza del giudice di pace ad irrogare una multa da 3.000 a 18.000 euro. Qui siamo all'aspetto umoristico: quale straniero

Inoltre la disposizione dell'allontanamento mediante accompagnamento in caso di violazione delle sanzioni è già stabilita dalla lettera *c)* del nuovo comma 4-*bis* dell'articolo 13 del testo unico,

conversione di un decreto‑legge, con questo tipo di atteggiamento rinunciamo, a prescindere, a svolgere il nostro ruolo di parlamentari, perché riteniamo che soltanto il Governo possa intervenire e, ove si possono portare contributi positivi, non vi accediamo?

quel briciolo di buon senso che, paradossalmente, si è manifestato proprio oggi in Commissione, dove ci siamo trovati a confrontarci su un atto del Governo che recepiva una proposta per il cambiamento dei visti dei cittadini dei Paesi terzi e abbiamo votato all'unanimità. Qualche volta dobbiamo interrogarci se, prescindendo un po' dalle categorie di maggioranza e opposizione, non si debba cercare di fare norme utili per i cittadini, tutti, e a prescindere dalle posizioni di parte.

Presidente, anche con l'emendamento 3.34 ritorno sul punto per dimostrare come, ancora una volta, rispetto ai temi del pericolo di fuga e alla possibilità di avere invece misure alternative al trattenimento nei CIE, noi abbiamo insistito in tutti i modi per migliorare questa norma alla Camera come al Senato. Rispetto al pericolo di fuga, che riguarda la non identità, il non possesso di documenti, la mancata possibilità di dimostrare che si ha un alloggio e altre condizioni, si aspetta la richiesta dello stesso immigrato, dello stesso soggetto che è su questo territorio, di chiedere la partenza volontaria e di farlo anche in un certo tempo. Questo tema è stato già illustrato da parte di altri colleghi, ma ci porta ad una contraddizione molto forte. Non avendo mai accolto nessuno di questi emendamenti e non avendo mai voluto modificare ed intervenire in qualche modo per utilizzare altre misure, voi finite con l'essere costretti a trattare tutta questa materia con il trattenimento nei CIE. Questo, oltre che essere una misura perniciosa e negativa dal punto di vista della restrizione delle libertà personali, si può intuire, non facilmente gestibile, sia per quanto riguarda la ricerca e la definizione delle identità - perché ingolferete le commissioni che dovranno fare questo lavoro sia per quanto riguarda i pericoli di ordine pubblico, di sovraffollamento e di possibile minaccia esterna che si verificheranno in determinate situazioni. Gli episodi che sono avvenuti sono all'ordine del giorno e ancora una volta ci ricordano che si potrebbero evitare situazioni situazioni peggiori in questo campo, se solo si volesse ascoltare e prendere in considerazione una serie di miglioramenti e di misure alternative.

che senza condizioni fossero ammessi i giornalisti all'interno dei CIE. Il passato di questa vicenda è abbastanza chiaro; il ministro Maroni ogni tanto sente il bisogno insopprimibile di mostrare i muscoli questo si è tradotto nel fatto che con circolari precedenti anche ai parlamentari è stato interdetto l'ingresso nei CIE. Alla senatrice Carloni è stato interdetto l'ingresso in un CIE ad aprile; all'onorevole Furio Colombo è all'onorevole Furio Colombo è stato interdetto l'ingresso in un CIE dopo telefonata diretta del ministro Maroni. All'onorevole Colombo è stato detto: «Se vuole, può venire domani»; mi sembra una risposta un po' provocatoria. Il problema della presenza dei parlamentari è stato - grazie al cielo - risolto, e abbiamo potuto constatare di persona quali sono le condizioni di alcuni CIE, su cui relazioneremo in altro contesto.

centri non servono nemmeno all'identificazione, perché si tratta per il 70 per cento di persone che sono state già identificate e che giacciono nell'inerzia più assoluta, perché non possono fare niente.

tutto ciò che il giornalista non vede la società ignora. È quindi fondamentale per noi che i giornalisti possano mettere occhi e mente in luoghi dove il potere politico vuole invece impedirlo.

che dovrebbero a nostro avviso rimanere in capo all'autorità giudiziaria. Siccome questo è uno dei punti che è stato anche oggetto di osservazioni, invito a votare a favore.

voto segreto,

Presidente, si accontentano di poco per entrare in euforia. Signor Ministro, faccio appello a lei personalmente, perché normalmente apprezzo il suo buon senso e la sua ragionevolezza, anche quando abbiamo opinioni politiche diverse e anche molto diverse.

quando risulta che nel caso concreto non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato

Per la durata di 18 mesi questa cifra vale qualcosa come 30.000 euro. Allora, mi chiedo, e le chiedo, signor Ministro, che senso ha quando con assoluta certezza, o ragionevole certezza, non c'è alcuna possibilità di procedere all'identificazione? Che senso ha tenere - e mi consenta - spendere in questo modo

il nostro emendamento tende puramente e semplicemente ad utilizzare in modo efficace delle risorse, per impedire il fenomeno dell'immigrazione clandestina, ma con politiche che non sono né barriere, né fazzoletti di qualunque colore messi sull'abito per mostrare una identità politica. La politica di contrasto all'immigrazione clandestina si fa in un modo serio ed efficace, e non con bandiere o con parole al vento. *(Applausi dal

sei mesi ad un anno e mezzo il tempo massimo di permanenza dello straniero nei centri di identificazione e di espulsione;

Il regime di libertà personale, all'interno di questa struttura, è sostanzialmente identico a quello della detenzione, con la differenza che ci troviamo di fronte ad una persona che allo stato dell'arte non ha commesso alcun reato. E lo stato di fermo, chiamiamolo così, è funzionale alla identificazione. Allora, crediamo che, poiché il numero dei centri di identificazione e di espulsione nel nostro territorio non è aumentato, e poiché semmai è aumentato - e le ragioni stanno nell'inefficienza dell'Amministrazione dell'interno, da un lato, e nella carenza degli accordi di cooperazione internazionale che sono funzionali alla collaborazione con gli Stati di provenienza ai fini della identificazione, la soluzione del problema non è allungare e addirittura triplicare il tempo di permanenza nei centri. La soluzione del problema sta nel rendere più efficiente il sistema che che porta all'accertamento della identità del cittadino straniero, nel rendere più efficienti i meccanismi attraverso cui si va all'accertamento dell'eventuale diritto alla protezione umanitaria e all'asilo, e certamente nel potenziare le relazioni internazionali che portano a far sì che le procedure di identificazione siano certe rispetto agli Stati di provenienza. L'idea invece di risolvere la questione nei termini prospettati dal Governo serve solo a serve solo a creare una situazione di disparità di trattamento, scaricando su queste persone un sistema di per sé inefficiente. Tutto ciò, con una serie di effetti paradossali, il primo dei quali è

con questa disposizione. Intendo dire che il tempo della custodia cautelare e della restrizione della libertà personale di cittadini italiani gravemente indiziati di gravi reati è è inferiore al tempo che noi prevediamo per la permanenza nei centri identificazione e di espulsione di soggetti la cui irregolarità non è stata accertata questo è il punto - e che quindi non hanno commesso alcun reato. Il secondo effetto di questa disposizione è che non si migliora il meccanismo, ma si intasano i centri di identificazione e di espulsione, perché è evidente che più tempo l'amministrazione ha a disposizione e più tempo impiegherà nel compiere gli adempimenti funzionali all'identificazione dei soggetti. Il terzo effetto è quello che, purtroppo, stiamo già vedendo

di costituzionalità della norma che abbiamo avuto modo di evidenziare nell'ambito della discussione sulla questione pregiudiziale, ci inducono a ritenere che si stia compiendo un gravissimo errore, che peraltro il Senato qualche mese fa,

un gravissimo errore, perché stiamo introducendo nell'ordinamento una norma che, da un lato, crea obiettivamente un'aberrazione dal punto di vista

Peraltro, stiamo anche lanciando un messaggio che obiettivamente non è dei migliori, perché ci mostriamo forti con i deboli, e allo straniero extracomunitario la cui dobbiamo accertare per capire se è un irregolare e quindi se va espulso diciamo che può stare in un sistema di privazione della libertà personale fino a 18 mesi; a chi invece si macchia di gravi delitti, con il nostro codice di procedura penale diciamo che può stare in carcere per un massimo di 12 mesi. Siamo garantisti a giorni alterni e lo siamo solo nei confronti di coloro i quali si trovano in una condizione di debolezza, mentre nei riguardi di chi si trova in una condizione di forza ci atteggiamo così come abbiamo fatto con il "processo lungo". Credo che sia obiettivamente vergognoso.

La seconda ombra lunga concerne la frequente violazione di diritti umani all'interno dei CIE, e si tratta, anche in questo caso, di un'ombra minacciosa sopra questa nostra istituzione. Una terza ombra lunga è di carattere giuridico.

per millenni, è stata abituata a considerare un comportamento normale? Nessuno vuole l'immigrazione irregolare, ma nella coscienza della gente l'irregolarità non è un grave reato, e allora non c'è proporzionalità della pena: credo pertanto che anche

il seguente: sappiamo che la probabilità di identificazione in un CIE tende a decrescere velocemente dopo le prime settimane. Dopo qualche settimana, addirittura dopo un paio di mesi, questa probabilità arriva arriva vicino allo zero. Ma allora quale razionalità c'è in una norma di questo tipo? Essa è assolutamente inconcepibile e, ripeto, irrazionale.

classificati secondo il momento di entrata. Vorrei sapere quanto tempo intercorre tra l'entrata nel CIE e il momento in cui viene fatta l'identificazione. Credo che allungando enormemente i tempi si aumentino i costi e si diminuisca enormemente l'efficienza. Infine, e non ultimo, chi viene trattenuto per mesi e mesi, anche per un anno e mezzo, in un CIE diventa inevitabilmente una bestia, e non può essere diversamente.

passati molti mesi, le condizioni di vita sono insostenibili, e tale situazione diventa poi il combustibile per quei conflitti e quelle rivolte nei CIE che rendono ulteriormente insopportabile la permanenza negli stessi. prego il Senato di riconsiderare questo allungamento, che è irrazionale sotto tutti i punti di vista e contrasta con i principi elementari di umanità, e credo anche del diritto, e quindi non va approvato.

o del Senato o bicamerale, sui CIE. Nel 2007 venne fatta una relazione da parte di una commissione indipendente presieduta dall'ambasciatore De Mistura, Mistura, che non ha avuto tempo di avere seguito ed è stata buttata nel dimenticatoio. Credo sia il momento di riaprire politicamente, seriamente e anche in maniera *bipartisan,* il *dossier* di questa istituzione, perché credo che tale

fino a 18 mesi nei centri di identificazione ed espulsione. Il carattere inumano di tali centri è già stato sottolineato da numerosi interventi precedenti.

e vengono a mancare anche le rare, insufficienti, miserabili prerogative di chi sta in carcere. Non c'è la possibilità di lavorare; non c'è la possibilità, entro certi limiti, di avere qualche momento di svago, se si può usare un termine così frivolo per una condizione così impossibile. È stato spiegato dai custodi di un CIE che non si può neanche tenere un biliardino, perché l'asse metallico divelto può diventare un'arma contundente. In definitiva, all'interno dei CIE i reclusi non possono fare nulla, ed è questo forse il motivo principale per cui, come ha spiegato il senatore Livi Bacci, l'uomo può diventare una bestia: perché non può esercitare nessuna prerogativa umana, ma può solo stare lì dentro; e trovandosi in tale condizione, nasce prima l'avvilimento e poi la rabbia. In secondo luogo, purtroppo, è testimoniato che, per lo meno per quello che riguarda i maschi, il 70 per cento dei detenuti dentro i CIE in realtà è già stato identificato, per cui si arriva all'assurdo che un centro di identificazione non riesce ad identificare gli identificati. Infine, devo ammettere un mio errore personale, e lo voglio sottolineare, anche se si tratta di una cosa considerata poco diplomatica. Nell'intervento precedente ho citato i casi della senatrice Carloni

ho trascurato di citare il fatto che il mio Capogruppo vuole che io non ricordi (invece lo voglio dire, perché gli errori devono essere ammessi in base al criterio della responsabilità personale) che il senatore Belisario è stato il primo

Io mi sono permesso di rielaborarli in un ordine del giorno al quale è stato dato parere negativo. Alcuni di questi impegni hanno invece ricevuto parere favorevole in altri ordini del giorno: ma tant'è.

limitare la durata massima del periodo di trattenimento e, in ogni caso, prevedere maggiori garanzie per le persone trattenute; prevedere un rilascio immediato di permesso di soggiorno nel caso in cui il trattenimento non sia giustificato anche per assenza di ragionevoli prospettive di allontanamento, come previsto dall'articolo 15, comma 4 della direttiva UE; non escludere dall'ambito di applicazione della normativa di recepimento la fattispecie dei respingimenti alla frontiera o differiti *ex* articolo 10 del Testo unico a prevedere la possibilità che nella valutazione delle singole posizioni sia possibile caso per caso rilasciare un permesso di soggiorno data la rilevanza umanitaria - ovvero la condizione psicofisica dell''interessato - di voler prendere in considerazione la richiesta avanzata; relativamente

presenze di migranti irregolari che spesso si trattengono nei territori dell'UE; e che tale risoluzione avverrebbe innanzitutto con un tentativo concreto di rimpatrio volontario assistito, mentre solo in casi in cui ciò non sia possibile si dovrebbe ricorrere ad un'espulsione forzata. Ricordando come sottoscritto anche dalla senatrice Carloni oltre che dai radicali, chiedeva di prendere ciò in considerazione una volta per tutte, ma non con termini particolarmente ordinatori e perentori. Ci è però stato detto di no, senza troppe spiegazioni. Vedo che

all'atteggiamento che si è avuto per adottare questo provvedimento relativamente alla direttiva. Pensiamo che questo atteggiamento produrrà di nuovo degli elementi di difficoltà per il nostro Paese.

arrestare gli immigrati e trattenerli in una situazione di carcere parallelo, non giustificato da alcuna

della disposizione in materia di trattenimento degli stranieri nei CIE, anche al fine di prevedere la riduzione del tempo massimo di trattenimento».

del diritto comunitario, perché voi avete scelto di recepire soltanto la parte più repressiva della direttiva in materia di rimpatri, mentre il suo nucleo fondante è quello di fare leva sul rimpatrio volontario ed assicurare una collaborazione anche con i Paesi di provenienza. Spero che il sottosegretario Mantica abbia l'accortezza di farsi carico di ciò anche nei confronti delle

a riferire semestralmente in Parlamento sull'utilizzo delle risorse dell'Unione europea destinate all'Italia per la gestione dei flussi migratori. Faccio veramente fatica a comprendere le ragioni per cui, visto che questo punto era già inserito nell'ordine del giorno

rispetto a quello che è stato illustrato dalla senatrice Fontana, nel quale peraltro si chiedeva semplicemente di fornire semestralmente un'informazione puntuale e dettagliata al Parlamento. Penso che ciò rientri nelle potestà del Parlamento: non vedo assolutamente cosa ci sia di male a tenere informate le Aule parlamentari su come vengono utilizzati questi fondi. Commissione, abbiamo approvato una norma in cui si chiede un aumento delle capacità operative a fronte della previsione di fondi e risorse nei confronti degli Stati membri maggiormente interessati dai flussi migratori. È giusto chiedere più fondi, ma è giusto anche che vi possa essere una forma di controllo da parte del Parlamento. Per questi motivi,

Signora Presidente, onorevoli colleghi,

richiede una particolare attenzione e senso di responsabilità da parte dell'Assemblea e di ciascuno

Polo:ApI-FLI)*. Stavo dicendo che il decreto-legge che oggi siamo chiamati a votare in quest'Aula richiede una particolare attenzione e un grande senso di responsabilità da parte di tutti noi. Per questo motivo, credo che i tempi di attenzione e di esame su questo provvedimento siano stati ancora una volta terribilmente strozzati, sia nell'esame in Commissione, sia oggi in quest'Aula. È stato detto, nel corso degli interventi sui singoli emendamenti, che sarebbe stato opportuno opportuno esaminare quali emendamenti non potevano essere accolti e quali invece avrebbero potuto migliorare questo testo che - come dicevo all'inizio - riguarda un problema

Le migrazioni, da sempre presenti nella storia dell'umanità, caratterizzano con connotati peculiari l'attuale fase storica di internazionalizzazione e globalizzazione. Negli ultimi vent'anni il fenomeno migratorio è stato caratterizzato da profondi mutamenti, parallelamente ai cambiamenti della società, che è entrata in un nuovo periodo di grande evoluzione. Questo insieme di fattori ha comportato un generale riassestamento della geografia e delle dinamiche delle migrazioni internazionali e una profonda modificazione dei cosiddetti *pull factors* e *push factors*. Va detto che i flussi migratori si pongono oggi con una incidenza tale da superare qualsiasi politica di contrasto e di restrizione adottata dagli Stati di destinazione. Infatti, accanto alla migrazione legale, assistiamo anche al sempre più vistoso ed esteso fenomeno della migrazione illegale che, per essere fronteggiato, necessita di un'appropriata disciplina, a livello nazionale ed internazionale, dei flussi migratori che tenti di conciliare le esigenze repressive dell'immigrazione clandestina con il rispetto dei diritti umani fondamentali internazionalmente sanciti e protetti. È, quindi, necessario fare una riflessione seria e matura sul fenomeno dell'immigrazione, mettendo da parte tutti i preconcetti e i pregiudizi - più simili ad una sterile propaganda politica - e affrontando in modo sereno ed equilibrato i vari aspetti che compongono il fenomeno dell'immigrazione.

con annunci che non si sono tradotti in iniziative concrete, volte ad arginare concretamente l'immigrazione clandestina. Continuiamo ad assistere ogni giorno a barconi di persone disperate che approdano nel nostro Paese. Che cosa è stato fatto? Sono state inserite misure sempre più restrittive, puntualmente bocciate dalla Corte di giustizia europea e che a nulla sono servite per ridimensionare un fenomeno al limite della tollerabilità. Serve una visione più ampia. Serve una prospettiva diversa. Serve un approccio maturo che porti ad interventi utili e concreti e non meramente propagandistici.

- che tutti sappiamo strozza il dibattito, circoscrive la discussione e impedisce (o per lo meno riduce ai minimi termini) qualsiasi contributo. dunque, si cerca, non di risolvere il problema, ma di rimandarlo. Viviamo in un'epoca in cui, più o meno inconsapevolmente, da più parti si tende a posporre la tutela dei fondamentali diritti civili ed umani

Da quest'ottica, la cittadinanza appare sempre di più determinata non tanto come *status*, ma come relazione tra il soggetto individuale e la comunità alla quale appartiene o della quale è venuto a far parte, accettandone le regole e condividendone i valori. E', quindi, necessario chiarire il concetto stesso di integrazione - di cui troppo spesso si parla senza capirne il vero significato - e da questo ripartire per creare una società basata sui doveri, ma anche sui diritti. Una vera integrazione può essere favorita da una nuova legge sulla cittadinanza, destinata ovviamente a quegli immigrati che si sentano realmente coinvolti nella vita della nostra società. Penso in particolare ai bambini, nati nel nostro Paese da genitori stranieri, che studiano nelle nostre scuole e per i quali occorre già da oggi preparare il loro futuro di nuovi italiani. Riguardo il cosiddetto decreto rimpatri, si è anche espresso l'Alto Commissariato ONU per i rifugiati, preoccupato per la tenuta delle norme in esame e determinato nel chiedere provvedimenti più miti per introdurre disposizioni più favorevoli alle persone interessate e nel rispetto degli obblighi internazionali sui diritti umani e sull'asilo. In particolare, l'aspetto più contestato del provvedimento riguarda il trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione sino ad un massimo di 18 mesi. Ovviamente, la previsione di siffatto trattenimento prolungato non è richiesta obbligatoriamente dalla direttiva rimpatri, ma è prevista come facoltà concessa agli Stati membri. sembra quindi che la previsione di questo ulteriore termine sia di natura meramente formale e serva a rassicurare l'opinione pubblica sulla volontà del Governo di assicurare una gestione rigorosa degli ingressi nel territorio nazionale. Tuttavia, lo stesso obiettivo potrebbe essere ragionevolmente raggiunto utilizzando un termine massimo di trattenimento ben inferiore a quello di 18 mesi, come quello previsto in via ordinaria dall'articolo 15, comma 5, della direttiva, e pari a sei mesi. D'altra parte, appare ben difficile che le situazioni che rendono possibile l'allontanamento si possano determinare a distanza di molto tempo dall'ingresso nei centri. Così come, oltretutto, la situazione di trattenimento, ove prolungato, potrebbe trasmodare in un sostanziale stato di detenzione per fatti non dotati di grande disvalore. Va ricordato che con il pacchetto sicurezza l'Italia aveva già aumentato questo periodo da due a sei mesi. Dalle statistiche dello stesso Viminale sappiamo che in pochissimi casi chi non può essere espulso in due mesi lo potrà in sei. Ora portarlo a 18 mesi è solo una punizione che non ha nulla a che vedere con una vera politica di rimpatrio, che non cambia l'effettività dell'allontanamento della persona dal territorio. È quindi solo un atto punitivo, viste le condizioni in cui versano questi centri.

L'estensione della durata massima di trattenimento nei CIE è ancora più preoccupante quando essa avvenga senza che siano previsti un rafforzamento delle garanzie e dei diritti dei soggetti trattenuti, né un adeguamento delle condizioni dei CIE stessi. sarebbe opportuno prevedere il rilascio immediato nel caso in cui il trattenimento non sia giustificato e in assenza di ragionevoli prospettive di eseguire l'allontanamento. Mi sento anche di dover sottolineare un aspetto di carattere generale. Si sta enucleando un diritto della cittadinanza europea applicato ai cittadini dell'Unione e ai cittadini extracomunitari. Le questioni sono complesse e mi rendo conto che sono anche difficili da risolvere tecnicamente. Mi pare che il Governo si sia mosso entro una cornice molto stretta: pur rispettando formalmente il dato europeo delle direttive, ne ha tuttavia accolto un'interpretazione eccessivamente estesa delle facoltà concesse agli Stati membri. Credo Credo che su tali questioni vada aperto un raccordo permanente con la Commissione europea che valga a prevenire l'insorgere di procedure di infrazione o peggio di sentenze come quella sulla clandestinità che sicuramente non rafforzano l'immagine italiana a livello europeo. infine, riguarda i minori cui l'articolo 17 della direttiva reca una disciplina specifica. Si dovrebbe rivolgere una grande attenzione a tale tema, perché i flussi di migranti comprendono un numero di minori e anche di donne veramente ragguardevole. Spero che si dia pronta attuazione anche a questa parte della direttiva, forse di scarso impatto nella prospettiva del rafforzamento del senso di sicurezza dei cittadini, ma di grande importanza nei confronti di categorie di persone estremamente vulnerabili, quali sono i minori. Quello che voglio dire è che serve serietà, tranquillità, buon senso e senso di responsabilità quando si trattano questi problemi, e serve anche più serietà quando si parla di vite umane.

Signora Presidente, colleghi, membri del Governo, signor Ministro, noi ci troviamo a pronunciarci su questo provvedimento, su cui annuncio il voto nettamente contrario del Gruppo dell'Italia dei Valori, in un momento che ci presenta alcuni esempi di vita recenti che sono molto espressivi. Ci sono i 25 immigrati rinchiusi dentro qualcosa che era il *pendant* della sala macchine di una barcaccia, gasati dagli effluvi venefici del motore acceso e ricacciati a colpi di bastone dentro il pertugio da cui cercavano di uscire, tutti allineati sul porto che li ha accolti, avviluppati nel telo di plastica. Questo è un esempio che sta fuori della nostra responsabilità: è avvenuto e lo constatiamo, ma fa parte del contesto. C'è un esempio invece che ci riguarda direttamente. Mi riferisco all'energumeno trevigiano che pensa di avere il diritto di spezzare la gamba all'immigrato senegalese solo perché costui non saprebbe rispondere alle domande in dialetto; brutta, bruttissima manifestazione di idiozia identitaria. Noi viviamo dentro questo mondo e votiamo oggi questo provvedimento con una procedura politicamente un po' curiosa. Molti colleghi, infatti, anche più avvertiti di me nella tattica della politica, hanno spiegato bene all'Aula il meccanismo con cui la cosa avviene è una sorta di voto di scambio tra l'approvazione da parte della Lega del «processo lunghissimo» che serve ad allontanare indefinitamente i processi al Presidente del Consiglio,

quando, come già molti colleghi e colleghe hanno detto, la procedura più saggia sarebbe quella di insistere invece con l'adozione dei criteri necessari per il rimpatrio volontario.

voglio rimarcare il fatto, non privo di significato, che la magistratura, che ha dovuto regolarsi di fronte ad un problema pressante, più volte e in più città, e in capoluoghi importanti (Firenze, Milano, Bologna, Venezia), ha adottato la direttiva europea direttamente, trascurando l'insufficiente legge italiana che non l'aveva ancora recepita, in base al criterio che il dettato delle leggi europee ha una prevalenza su quelle italiane. Il comportamento dei magistrati che hanno fatto questo è educativo: serve a capire che, di fronte ad un tema dolente, l'adozione del punto di vista più avanzato permette di fare meno errori. Uno dei motivi pressanti per cui non si può accettare questo provvedimento è la forzatura retorica che viene fatta del limite dei 18 mesi. Questi 18 mesi stanno nella delibera europea, ma se si va a vedere tale delibera si scopre che quei 18 mesi sono un termine praticamente irraggiungibile, perché è pensabile soltanto in determinate condizioni particolarmente difficili e subcondizioni altrettanto particolarmente difficili.

della severità repressiva a confronto della dolcezza di quelli che non sanno fare niente, cioè il centrosinistra. In realtà, il Senato aveva già approvato, all'incirca all'incirca un anno fa, una norma in cui questo limite era di sei mesi e non si capisce perché oggi dovremmo adottare in senso forzoso il limite di 18 mesi quando ci siamo già dati una regola più restrittiva che è faticoso applicare perché, come anche altri senatori hanno rilevato, o l'identificazione avviene nel primo periodo di detenzione dentro questi centri oppure la possibilità dell'effettiva identificazione si allontana e svanisce. Già sei mesi è un tempo lunghissimo, è quasi il tempo di una gestazione: non è immaginabile che si possa prolungare a dismisura la detenzione in luoghi che sono luoghi di inedia. Due parole su questo. La condizione di chi è recluso in questi Centri di identificazione ed espulsione è veramente anomala, è come in un limbo *extra* legale: non è carcere e non è società. Non ha né i vantaggi della società, né le prerogative elementari formali del carcere; è una specie di terra di nessuno che da parte del potere politico si cerca di contrabbandare come addolcita dalla presenza di organismi di aiuto, di strutture di sostegno, di volontariato attivo e così via, che ci sono sicuramente. Sono pronto ad ammettere che molti CIE non siano *lager* veri e propri, nel senso dell'esercizio della pura brutalità. Ma facciamone anche esclusione completamente e immaginiamo che nessun CIE sia un luogo di materializzazione della pura brutalità. Che cosa resta? Resta qualcosa di terribile che ripugna alla coscienza civica: resta un luogo dove non esiste libertà alcuna di esercitare alcuna attività umana che non sia quella della pura sopravvivenza. Questo corrisponde all'inedia forzosa e coatta, che genera, come si diceva, prima avvilimento e poi rabbia. E c'è l'altra contraddizione immanente dei Centri di identificazione e di espulsione, su cui voglio tornare per un secondo. per cento dei maschi reclusi in questi Centri, si tratta di persone già identificate, che hanno già avuto esperienze carcerarie, che sono state condannate, che hanno addirittura scontato la pena. Come si fa a dire che questi non sono identificati? Questi sono identificati, ma i centri di identificazione non lo fanno. Qual è la via di fuga salvifica di questa ignoranza? È il fatto che gli Stati di provenienza si rifiutano di riconoscere provenienza nazionale e nota anagrafica. Ma si può attribuire la responsabilità della inazione degli Stati ai poveracci che sono in quel momento detenuti e che non hanno nessuna responsabilità di questa inazione? Qui siamo di fronte ad una dislocazione della responsabilità che ha qualcosa di terribile. Lo Stato di provenienza non opera secondo giustizia ed il soggetto proveniente dallo Stato di provenienza ne paga le spese. E ne paga le spese, tra l'altro, secondo un meccanismo di indeterminatezza che - mi passi il paragone dal punto di vista strutturale - ha qualcosa a che vedere con Guantanamo. Guantanamo è un luogo di brutalità, di coercizione e di torture. Per carità, queste cose non ci sono, sono, ma fondamentale è lo stato di incertezza, il non sapere. Penso che la questione dell'immigrazione sia troppo vasta e troppo tesa per affidarla a soluzioni di tipo repressivo. Il ministro Maroni è occupato con le sue comunicazioni. Ma vorrei che la Sottosegretaria che sta ascoltando, sommessamente ripetesse al ministro Maroni un suggerimento di lettura. Consiglio due letture di due diverse epoche: la prima, il volume «Sull'Oceano» di De Amicis

È un volume intero che racconta l'esperienza a bordo di una nave, dove minutamente si vede il brulicare di umanità degli italiani che vanno a fare gli emigranti in Argentina. Suggerisco poi

ad una dimensione repressiva. Per finire, signora Presidente, bisogna puntare sui rimpatri volontari ed anche su quello che c'è di buono che viene dall'immigrazione. è una proposta che ha come capofila l'ARCI, che è un disegno di legge di iniziativa popolare che punta a dare il voto amministrativo agli immigrati che hanno un radicamento reale. In due parole, chi lavora e chi manda i figli a scuola ha diritto di voto ha diritto di voto nel nostro Paese, se non altro, per lo meno sul piano amministrativo. In questa maniera, possiamo accogliere il contributo vitale di persone che vogliono e possono continuare ad abitare e a lavorare, e anche a migliorare e a migliorarci,

affrontando in questo modo e in tutta fretta il problema dell'immigrazione? Sia ben chiaro: noi siamo assolutamente contrari all'immigrazione clandestina,

L'unica speranza è che questo provvedimento presto sarà dichiarato incostituzionale. Esso, però, è sbagliato anche nella sostanza perché, oltre a presentare anch'essa indubbi profili di incostituzionalità, come evidenziato nella nostra questione pregiudiziale di stamani, tenta di affrontare materie delicatissime come l'immigrazione e il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi irregolari in un'ottica emergenziale, anziché in una visione finalmente di lungo periodo. Non solo, la confusione che talvolta regna in quest'Aula e l'indifferenza dinanzi all'esame di provvedimenti così importanti, che comunque devono - lo sottolineo non sempre fanno conoscere in modo adeguato ciò di cui si discute. Avrei il desiderio di parlare con ciascun parlamentare della maggioranza per chiedere a ognuno se realmente ha approfondito il problema di un individuo che, solo perché di colore di pelle viene messo in un centro di identificazione per un anno e mezzo senza aver commesso alcun reato.

ma veramente si pensa che al termine dell'anno e mezzo succeda qualcosa, se non un foglio, messo in mano all'immigrato da parte del prefetto, in cui si dice a costui che deve lasciare il nostro Paese? L'unica differenza è che costui si è trasformato in una iena, perché un anno e mezzo di centro di identificazione lascia segni indelebili su qualunque essere umano!

non c'è una valutazione della sussistenza di un quadro indiziario e cautelare sufficiente, e soprattutto i termini di durata della misura superano di gran lunga quelli fissati dal codice di procedura penale e appaiono assolutamente sproporzionati rispetto al risultato che si vuole raggiungere. Il Ministro sa quanta stima ho per lui e per la sua saggezza, ma mi chiedo come abbia potuto avallare 18 mesi di carcerazione, laddove l'articolo 303 del codice di procedura penale fissa ben altri termini termini e tempi per coloro che un reato sono sospettati di averlo commesso realmente. Se io ho ucciso una persona non posso stare preventivamente in carcere più di un anno:

Non sarebbe meglio mettere in atto politiche che diano spazio a seri accordi bilaterali preventivi con Paesi terzi piuttosto che ricorrere a tempi così lunghi, trattenendo chi non è colpevole di alcun reato? Non sarebbe meglio puntare piuttosto su un lavoro stretto, costante e coordinato tra tutte le polizie? Siamo ben coscienti che, se uno straniero non viene identificato subito - in un mese, in due mesi, in tre mesi? - non lo sarà più. non lo sarà più. Parliamo chiaramente, si pensa di dilatare il tempo di detenzione solo per scoraggiare gli arrivi dei migranti, ma questa non è la politica giusta: così non si affronta seriamente il problema migratorio. Senza dimenticare poi i costi che i centri comportano, e soprattutto senza affrontare il tema fondamentale delle condizioni in cui i migranti sono costretti a vivere in tali strutture, rispetto alle quali l'Alto Commissario per i rifugiati ha chiesto al Parlamento un rafforzamento delle garanzie e dei diritti dei soggetti trattenuti. Non condividiamo di certo le violenze perpetrate ieri dagli immigrati del CIE di Bari; le condanneremo sempre, e sosterremo sempre le forze dell'ordine - soprattutto quando ad intervenire è il sottoscritto - ma non si può non comprendere il perché centinaia di immigrati blocchino strade e binari per protestare contro il ritardo

Ribellione, scontri, feriti: è ciò che si ottiene da una politica come questa. Voglio sottolinearlo ancora una volta: siamo di fronte all'ennesima conferma

esimo dal definire l'ultimo provvedimento sulla giustizia - e tu mi regali un decreto come questo, finalizzato unicamente alla gente di Pontida, quella della: «Secessione! Secessione!». Respingimenti utilizzati ormai come *spot* e propagandati in provvedimenti come quello oggi al nostro esame. Governare l'immigrazione non significa mai seminare paura tra la gente, come ormai è abituato a fare questo Governo fin dal primo giorno della campagna elettorale. Questa politica non fermerà certo gli arrivi, né gli sbarchi, che, voglio ricordarlo al di là di ogni propaganda, rappresentano solo la minima parte del problema migratorio. Questa politica non fermerà le stragi del mare, come quella dei 25 migranti morti soffocati in un barcone. Che dire poi dei problemi relativi ai minori, anch'essi trascurati da questo testo? Così come la questione dei figli degli immigrati, che richiama a sua volta un tema che il Parlamento avrebbe dovuto da tempo affrontare, cioè quello della cittadinanza, dello *ius soli* rispetto allo *ius sanguinis*, oltre ai complessi problemi di immigrazione che riguardano i migranti. Ci rendiamo conto che non è concepibile in alcun modo che non si preveda una soluzione per l'acquisizione della cittadinanza in modo più snello per i minori stranieri nati nel nostro Paese? In relazione poi ai provvedimenti di espulsione, se è condivisibile il passaggio relativo alla partenza volontaria, non vi è alcun accenno all'obbligo di valutare il rispetto del principio di non respingimento e dei divieti di allontanamento per i per i richiedenti asilo e protezione internazionale. Sembra ci si dimentichi poi del presupposto fondamentale: la migrazione è spesso generata da veri e propri drammi umani ed è figlia della povertà e della disperazione. e della disperazione. Ecco allora che l'azione politica dovrebbe consistere anzitutto nel riconoscimento ai migranti del nostro Paese del medesimo rispetto che dobbiamo a noi stessi. Il pretesto di ottemperare a obblighi internazionali non può spingerci a convertire un decreto controproducente. Per ognuna di queste ragioni esprimiamo con sofferenza una posizione negativa. Avremmo voluto dare un giudizio diverso,

Signora Presidente, colleghi senatori, signori Ministri e Sottosegretari, pare che in alcune canoniche circostanze una parte politica, di centrosinistra, non possa fare a meno di rovesciarci, e rovesciarsi, addosso un copioso profluvio di frasi fatte*, slogan*, rituali e approssimative sentenze, caro senatore Serra. Ne riceviamo ulteriori conferme trattando della gestione degli ingressi stranieri, argomento che suscita riflessi condizionati, come il martelletto del dottore sul ginocchio del paziente. Lo stimolo, in questo caso, deriva dal recepimento da parte del Governo italiano di due direttive comunitarie, dei cui testi ci sentiamo di raccomandare la lettura integrale. Tale semplice ma prezioso accorgimento avrebbe forse suggerito una maggiore continenza verbale, a partire da quel carosello di spauracchi agitati in questi giorni da esponenti politici o politicizzati. E davvero, colpisce che, contestualmente al varo della normativa originata dalle due direttive, si sia alimentato financo un movimento di pressione che ha per sigla il gioco di parole «LasciateCie entrare», che invoca - l'hanno ricordato tanti interventi dei senatori dell'opposizione quest'oggi - il libero ingresso dei giornalisti nei centri di identificazione ed espulsione, il tutto in nome della Costituzione, o meglio di quell'articolo 21 il quale in verità attribuisce e proibisce le censure preventive e reprime le pubblicazioni contrarie al buon costume, ma non fa cenno della circostanza in oggetto.

Lo consiglio caldamente pure al capogruppo dell'Italia dei Valori, senatore Felice Belisario, che, dopo avere tirato in ballo i *lager*, ha definito in varie occasioni carceri a cielo aperto i CIE di tutta Italia. Ebbene, se il senatore Belisario, dall'esperienza infelice di quest'oggi sul voto segreto, avesse letto la direttiva comunitaria, non troverebbe nulla di nazista, ma tutto di europeo nella sua similitudine tra carceri e Centri di identificazione ed espulsione. direttiva infatti viene specificato che il trattenimento dei clandestini può avvenire negli appositi CIE o,

è quanto consente l'Europa, ed è ciò che tuttavia il nostro Governo non si spinge a prescrivere, preferendo per zelo umanitario disporre la collocazione degli immigrati irregolari in luoghi diversi dal carcere. Ai sindacalisti della Federazione nazionale della stampa, impegnati nella campagna per il libero ingresso dei giornalisti nei CIE, verrebbe così da domandare: a quanti di loro e dei loro colleghi, e dove, è mai consentito il viavai in prigioni e luoghi affini? E tuttavia, qualora il Ministro lo giudicasse opportuno, ovvero congruo avuto riguardo alle primarie esigenze di sicurezza dei luoghi e di riservatezza delle persone ivi trattenute, penso che la stessa istanza dei sindacalisti della stampa potrebbe trovare accoglimento, nei modi e con le garanzie dovuti. Che dire poi del preteso scandalo costituito dai paletti alla libera circolazione di cittadini europei sul suolo comunitario? Tutto scritto e sancito proprio da Bruxelles all'articolo 27 della direttiva, dove si stabilisce che gli Stati membri possono limitare la libertà di circolazione di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica. È un principio recepito dalla normativa nazionale in oggetto, la quale specifica come a carico dello straniero comunitario da allontanare debbano riscontrarsi comportamenti che costituiscono minaccia concreta effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. Forse queste misure suscitano tanta avversione in certa parte politica perché vengono mentalmente associate alle richieste di cui il nostro movimento, la Lega Nord, non da oggi, si fa portatore. Ragioniamo semmai sul fatto che tali istanze appartengono non solo alla deprecata cultura leghista, bensì alla cultura giuridica e sociale dei Paesi europei. Entriamo finalmente nel capitolo dei fatidici rimpatri, che suscita la veemente riprovazione di quanti vagheggiano ingressi liberi e assistiti. Buonsenso oggettivo, premura verso la propria gente e onestà intellettuale nei confronti di chi nutre fuorviate attese motivano gli allontanamenti dal suolo nazionale di immigrati privi dei requisiti richiesti. La circostanza risulta all'articolo 3 della direttiva, con tanto di nulla osta al rimpatrio di cittadino di Paese terzo, specificando che ciò avviene sia in adempimento volontario di un obbligo di rimpatrio sia forzatamente. Il decreto del Governo provvede al perfezionamento degli strumenti atti a tale scopo, riconosciuti come convenienti in sede comunitaria, adattandoli alle esigenze reali. Tra questi, è emersa l'opportunità di procrastinare sino a 180 giorni il trattenimento degli immigrati irregolari, pietra dello scandalo nella discussione di oggi. Ebbene, tra quanti spacciano questa misura come una sorta di arbitraria detenzione di sei mesi, qualcuno si è preoccupato di specificare che ordinariamente la permanenza nei centro di identificazione Che la proroga successiva di un altro mese motivata da gravi difficoltà d'identificazione sarà richiesta e ottenuta dal questore presso il giudice? Che tale meccanismo di garanzia verrà ulteriormente applicato alle proroghe successive? E che, ultima domanda, il prolungamento il prolungamento della permanenza non può addebitarsi a malevolenza di legislatori, tutori dell'ordine e magistrati, bensì al rifiuto opposto dal clandestino nel fornire elementi atti alla propria identificazione? Mi rammarico, e concludo, che sui temi dell'immigrazione risulti sempre faticoso sfrondare la discussione dagli artifizi della propaganda. Noi crediamo di aver guardato la sostanza delle proposte normative in esame; ne abbiamo maturato la nostra valutazione positiva riconoscendone l'idoneità a coniugare l'efficacia nell'azione dello Stato e un valido patrimonio di garanzie. diritti che condividiamo, al pari dell'intero provvedimento, perché attribuiti a soggetti deboli, che una cinica demagogia riduce spesso a vittime di ingannevoli aspettative.

Presidente, colleghi, Ministro, rappresentanti del Governo, cercherò di illustrare le tre ragioni fondamentali per le quali il Gruppo del Partito Democratico voterà contro questo provvedimento, che pure è in applicazione di due direttive dell'Unione Europea, per una delle quali siamo già in procedura d'infrazione, mentre per l'altra siamo ai prodromi della procedura. È, quindi, giusto che il Parlamento si preoccupi di recepire la direttiva; ciò nonostante voteremo contro, per le ragioni che cercherò di esporre, con qualche difficoltà che mi deriva dal suo silenzio, perché non ha voluto replicare al dibattito che c'è stato questa mattina. Se non per rispetto nei nostri confronti, poteva almeno cogliere l'occasione per dire due parole di cordoglio per i 25 morti di ieri - queste parole le abbiamo sentite pronunciare solo dal presidente Chiti - vittime della tratta spietata di esseri umani, e per informare l'Aula dei gravi disordini avvenuti in Puglia, una vera e propria rivolta,

incidenti, non ritiene sia il caso di parlarne oggi, mentre stiamo per votare questo provvedimento; infatti, parlarne significherebbe leggere la realtà e

perché certificherebbe il fallimento della politica sull'immigrazione. Si tratta di una politica costituita da misure restrittive e da una logica puramente securitaria, che non aiuta le espulsioni e crea situazioni di enorme di cui sono vittime innanzi tutto gli stranieri extracomunitari, ma anche le comunità locali. Altri colleghi hanno già ricordato la polemica sorta quando non sono state prese in considerazione le nostre proposte per piccoli centri disseminati,

è riesaminato ad intervalli ragionevoli su richiesta del cittadino di un Paese terzo interessato o d'ufficio. Nel caso di periodi di trattenimento prolungati il riesame è sottoposto al controllo di un'autorità giudiziaria». Noi cioè non

si dice: «La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli alle persone cui si applica, purché compatibili con le norme in essa stabilite».

non serve a nulla tenere le persone nei CIE, o in carcere, e, se non si riuscirà a identificarle nel giro di due o tre mesi non sarò più aiutarli invece a rendere possibili le espulsioni, a renderle praticabili, effettive, perché, già prima delle vostre leggi, tra i procedimenti assunti e quelli effettivamente

mettete rimedio alla magistratura cattiva, all'Europa cattiva (come se il nostro Commissario fosse stato addormentato quando si sono votate certe cose) che

Vengo ora alla seconda ragione, quella che riguarda l'efficacia e la gestibilità delle norme, e non la propaganda. Qui non si tratta di essere buonisti o cattivisti: sicuramente non bisogna essere propagandisti. Con i rimpatri volontari fatti così, con le norme qui introdotte, noi rendiamo tutto complicato - come abbiamo cercato di spiegare in tutti gli interventi - mentre noi dovremmo favorire al massimo, supportare,

caro Ministro, lei e i suoi colleghi avete fatto un decalogo di richieste. Per adesso abbiamo visto tre uffici che hanno rubato spazio ad un Istituto d'arte che era ospitato nella Villa Reale di Monza. Tre uffici su cui avete scritto: «Ministero della semplificazione e Ministero

che rendono inapplicabili - e quindi si prende in giro la gente - le misure cosiddette securitarie, e

Sono state utilizzate definizioni del provvedimento che a ben vedere non solo non hanno ragione di essere espresse in questi termini, ma che non corrispondono minimamente alla realtà. Sostenere per esempio che l'internamento nei CIE equivale ad una condizione peggiore rispetto alla carcerazione significa non dire la verità. Possiamo aggiungere che questi provvedimenti sono, per fortuna, non per volontà della maggioranza o dell'opposizione, assistiti da garanzie fondamentali, che trovano nell'articolo 13 della Costituzione, per cui la libertà personale è inviolabile e può essere compressa solo nei casi previsti dalla legge, con provvedimento motivato dell'autorità giurisdizionale Mi piace ricordare qui una famosa definizione di Ortega y Gasset: l'uomo non ha natura ma ha una storia. E la storia dell'uomo è quella dei diritti fondamentali e umani, che qui sono stati dichiarati calpestati

alla sicurezza dei cittadini. Sin dalla Dichiarazione del 1789, la libertà è accompagnata anche e sempre dalla sicurezza. Nel secondo emendamento della Costituzione più antica del mondo, quella degli Stati Uniti, si parla di libertà e sicurezza. Nella Carta dei diritti fondamentali si parla di libertà e sicurezza. La sicurezza, quindi, è l'esigenza di garantire i diritti fondamentali, appunto, dall'oppressione, dalla criminalità. E non vi è dubbio che nelle maglie dell'immigrazione irregolare vi siano sacche di criminalità, o comunque di pericolosità.

Allora, forse è giunto il momento di chiederci se queste misure, che non sono certamente lesive dei principi e dei diritti di *habeas corpus*, ledono il principio fondamentale inviolabile della dignità di queste persone nei CIE. CIE. Quindi ritengo che l'accesso dei parlamentari e delle associazioni possa far evidenziare tutto questo, ma nessuno può affermare che all'interno di questi istituti ci siano delle compressioni dei diritti fondamentali dei cittadini. Qualcuno ha qui sostenuto la tesi che questo provvedimento viene approvato in luogo di uno scambio politico: processo lungo in cambio delle espulsioni; non è così. Naturalmente non è questa la sede per discutere dei temi che abbiamo trattato qualche giorno fa, ma vorrei ricordare che il principio di escutere i testimoni a difesa non solo trova fondamento nell'articolo 111 della Costituzione, ma principalmente nell'articolo 24, che contempla il diritto di difendersi provando la propria innocenza. Queste frasi sono di un partigiano, di un uomo di diritto, di un ex presidente della Corte costituzionale, Giuliano Vassalli, che prima della modifica dell'articolo 111 della Costituzione aveva già enucleato questo principio fondamentale di un processo di parti in cui il diritto di escutere i testimoni corrisponde al *Right to Examination* del diritto processuale accusatorio anglosassone. Certo, si può discutere sulle misure che oggi il nostro Paese appronta per assicurare l'identificazione degli stranieri, posto che nessuno può porre in dubbio che uno Stato abbia il diritto di identificare chi vive nel territorio nazionale privo di identità e privo di documenti di identificazione, ma vale la pena ricordare che queste norme si applicano secondo il principio di frammentarietà, nel senso che le forze di polizia accompagnano nei centri di espulsione quei soggetti che, secondo circostanze di tempo e di luogo, possono apparire pericolose per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. E le ragioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica costituiscono il fondamento per l'adozione dei provvedimenti di espulsione. nel nostro diritto (quindi invito tutti a valutare e a leggere queste norme con gli occhiali del giurista, come diceva Jemolo, e non certo con gli occhiali e la vista della contrapposizione politica), nell'applicazione di queste norme, siano perfettamente compatibili alcune cause di giustificazione, quella nuova, «salvo giustificato motivo», o quella preesistente dello stato di necessità. Il nostro quindi è un sistema e uno Stato di diritto in cui i diritti fondamentali sono garantiti a livello costituzionale da una giurisdizione piena e consapevole delle sue funzioni e delle sue garanzie fondamentali, ma vorrei richiamare anche la funzione fondamentale, importante, che la Suprema Corte di cassazione assicura in base agli articoli 606 e 607 del codice di procedura penale alla corretta applicazione del diritto e alla corretta applicazione della giurisprudenza. Quindi, conclusivamente, signora Presidente e onorevoli colleghi, vorrei aggiungere che questi provvedimenti non possono essere il fomite per comprimere il nostro Paese o per farlo passare per un Paese incivile, perché credo che l'Italia abbia tutti i requisiti e le caratteristiche per far sì che la nostra sia una vera democrazia, basata sullo Stato di diritto e con piena divisione dei poteri. Il Governo ha portato in quest'Aula del Parlamento il provvedimento che oggi ci accingiamo a votare. Il Gruppo del Popolo della Libertà lo vota convintamente, certo che le garanzie sistematiche e costituzionali che esistono all'interno della nostra democrazia e all'esterno, tramite la Corte europea dei diritti dell'uomo, sapranno garantire a tutti certezza del diritto, garanzia di libertà e, soprattutto, sicurezza ai cittadini onesti contro la criminalità. *(Applausi

colleghi, vi prego, non mi costringete a sospendere la seduta per questo baccano. Chi deve lo faccia, possibilmente in silenzio, e consenta al senatore Grillo e a noi tutti di procedere nei nostri lavori. Signora Presidente, utilizzo i pochi minuti a mia disposizione per illustrare i motivi in forza dei quali ho presentato l'ordine del giorno G2, nel quale si ipotizza un processo di razionalizzazione dei servizi e delle strutture attualmente organizzate nel Senato della Repubblica. L'idea di questo ordine del giorno di far sì che il Consiglio di Presidenza del Senato possa prendere quanto prima accordi con la Camera dei deputati affinché si possano assieme gestire alcuni servizi in comune. Ritengo che un processo di razionalizzazione in questo senso

Chi rimane consenta a tutti di seguire. Altrimenti, esistono sale accanto. GRILLO

agire su questo versante, facendo esperienza dei risultati positivi di alcuni istituti introdotti - ad esempio, lo strumento del *global service* - per ottenere maggiore efficienza organizzativa e un contenimento dei costi. L'idea fondamentalmente è quella di unificare alcuni Servizi e Uffici. Faccio un esempio: gli Uffici stampa di Camera e Senato, a mio modo di vedere, potrebbero essere unificati, così come potrebbero essere unificati alcuni Servizi che

e il Servizio informatica. L'unificazione di questi Servizi e di questi Uffici porterebbe automaticamente ad una razionalizzazione degli stessi e ad un contenimento delle spese.

che potranno esserci resistenze degli apparati interni, ma se siamo obbligati a realizzare contenimenti nei costi di gestione, se siamo obbligati a razionalizzare la spesa, se siamo obbligati a fare tutto quello che farebbero nelle nostre condizioni imprese private per realizzare economie di gestione, non vedo come si possa rinunciarvi

nei prossimi mesi: è un processo che va avviato, ma credo che nel medio termine potremo portare a casa questo risultato. Questo anche nella prospettiva di una riforma costituzionale, di un Senato che svolga funzioni diverse da quelle che finora ha svolto. Faccio presente da ultimo, signora Presidente, che parliamo di questa idea, di questa razionalizzazione e di questa riforma dei Servizi e della struttura ormai da più di dieci anni, ma evidentemente finora non c'è stata una forte

hanno una caratterizzazione quasi surreale, aggettivazione che è stata utilizzata ben poco dai colleghi intervenuti, che a mio avviso si sono ristretti, nel loro parlare, molto più a discorsi che riguardavano la perimetrazione propria, matematico-finanziaria del bilancio, piuttosto che considerazioni che afferiscono ai presupposti della formazione o, con un parlare forse presuntuosamente forbito, alla filosofia che viene posta a base della redazione del bilancio, che poi è la riclassificazione e l'evidenziazione della vita del Senato e, unitamente a quella della Camera, della vita del Parlamento italiano. Perché faccio questa premessa? Perché nell'intervenire all'interno del perimetro mi è sembrato tanto di vedere un gruppo di medici che si fossero messi a parlare di quale unguento utilizzare sull'esantema di una malattia quale il morbillo, la scarlattina o la rosolia, non rendendosi conto che non è una semplice orticaria ma una malattia molto grave; o, parlando in termini bellici, è come se, ripercorrendo la storia della Seconda guerra mondiale, si dicesse che il bombardamento degli armamenti era una cosa inutile e invece bisognava rispondere allo schieramento di forze con altro schieramento di forze. Perché dico questo? Perché alla ipocrisia e alla demagogia con la quale si fa lievitare l'antipolitica in Italia si risponde con una difesa che nulla di ragionato e che non cerca di evidenziare e sviscerare quelli che sono i presupposti dell'antipolitica. E perché questi presupposti sono l'antipatia, l'astio del popolo italiano per quello che il Parlamento, espressione del popolo, non fa. Se oggi ponessimo una domanda all'italiano medio su qual è l'indennità da pagare

ci direbbero che noi non dovremmo essere pagati, così come faremmo noi se fossimo gli azionisti di un'azienda che invece di produrre utili costruisce perdite, perché questo Parlamento, la politica italiana, per le speranze, per le aspettative degli italiani è un consiglio di amministrazione che non dà alcuna risposta, che produce ancor più vessazione e ancor più tassazione, che produce ancor più frustrazione rispetto a quelle che sono le aspettative per noi e per i nostri figli. il parlamentare medio che non vede il proprio figlio avere aspettative che vengono coronate all'estero? Perché le famiglie

il contenimento dei costi della politica, con quella che a nostro avviso, modestamente, era stata individuata come una violazione costituzionale. Infatti, ricordo ai colleghi la Costituzione prevede che l'indennità deve essere fissata dalla legge. Il Governo degli italiani invece ha voluto proporre che questa indennità non venisse fissata da una legge italiana, perché, se quell'articolo fosse rimasto così com'era stato proposto, tale indennità avrebbe dovuto essere fissata da una decisione legislativa del Parlamento della Lituania o del Parlamento della Serbia, perché, quando si parla di media delle indennità dei Paesi UE, questo significa che noi, alla faccia dello sciovinismo preteso (che poi forse lo potremmo chiamare brambillismo, perché magari in Francia hanno Chauvin e noi finiamo soltanto per avere Brambilla, e quindi il brambillismo, e non è cosa opportuna), avremmo delegato, secondo quel ragionamento, la fissazione della nostra indennità - e quindi non il costo, ma la vita della democrazia, perché la vita della democrazia si consustanzia nella vita del Parlamento e nella delega che il cittadino dà al suo eletto - alla eletto - alla decisione del Parlamento della Lituania. Oggi invece abbiamo un po' rimediato: deleghiamo questa decisione alla decisione del Parlamento francese, tedesco (e ancora qui passi), ma anche del Parlamento portoghese, di quello spagnolo e di quello belga. Ma vi rendete a che punto siamo arrivati? A parlare dell'unguento sull'esantema o, del pannicello caldo, invece di parlare del perché c'è l'antipolitica. C'è l'antipolitica perché questo Paese si è trasformato, ha materializzato - come dicono i costituzionalisti - la scelta di un Governo e non ha materializzato l'attività del Parlamento. Dopodiché, nessuno di voi, nessuno di noi ha avuto il coraggio di formalizzare quella materializzazione. Si pensi a quello che in Francia è avvenuto dopo che con De Gaulle il gollismo si credeva dovesse finire, e invece le istituzioni sono state capaci di reggere alla fine di De Gaulle, talché è continuata la fase della Quinta Repubblica. Noi invece non facendo questo cosa abbiamo? Abbiamo un Parlamento che non ha la capacità, per la vostra manchevolezza (e mi rivolgo ai colleghi dell'altra parte dell'emiciclo) e per la vostra incapacità di essere propositivi rispetto a una trasformazione non soltanto materiale ma profondamente formale, di dare una risposta ai cittadini e balbettiamo di leggi elettorali non rendendoci conto che prima c'era la carta moneta, mentre oggi c'è tanta di quella moneta per cui sarà possibile - e dobbiamo sperare che non lo sia - che di monetine ce ne saranno a disposizione per tutti. Questo, infatti rischiamo che succeda: rischiamo di essere travolti dall'antipolitica. E quando pensiamo che certi giornali scrivono queste cose perché sono perché sono alimentati, indirizzati, suggeriti, non ci rendiamo conto che invece i libri, come quelli sulla casta, non vengono letti perché qualcuno venga forzato a comprarli, ma perché i nostri parenti, mia zia Iolanda, la cugina della mia mamma o l'amica di mia moglie finiscono per comprarlo e per domandarci con un sorrisino quanto è il nostro guadagno; e quello che leggono non è quanto prendiamo, non è l'indennità, ma di quanto la diminuiamo: allora fanno il ragionamento che se la diminuiamo di 1.000 euro, chissà di quanto è l'indennità. E nulla si fa in questo Paese, nulla fa il Governo; anzi, nulla facciamo noi: perché dire il Governo, perché dire i Questori, perché dire la Presidenza del Senato o la Presidenza della Camera? Nulla facciamo noi per ergerci a difensori della nostra dignità. *(Applausi dal Gruppo* *PdL).* Nulla facciamo noi per dire che il vitalizio è un istituto giuridico completamente diverso dal trattamento di quiescenza, che è garanzia di democrazia e che, visto che ci sono i diritti quesiti (come si ricorda negli ordini del giorno presentati da tutti) non avremo nessuna preoccupazione per quello che è il nostro diritto. Ma la nostra preoccupazione è per il diritto di quelli che verranno, perché, se continuiamo con questo andazzo, a voler fare i parlamentari penseranno soltanto coloro Non pensiamo e nessuno ragiona sul fatto che questo attacco che oggi altri colleghi hanno lanciato nell'altro ramo del Parlamento non è un attacco al vitalizio: è un attacco alla democrazia e alla garanzia della democrazia che noi tutti impropriamente, al di là dei

hanno la possibilità di rinunziare a quest'indennità perché sono magistrati? Quanti magistrati non rinunziano alla loro indennità, che è più alta della nostra, e continuano a prenderla, facendo

Se in letteratura in altri casi viene detto che quando certi ragionamenti sono fatti con fervore possono essere, se riguardano la gioventù, la febbre la febbre della ragione; credo che invece la nostra senilità (e ancor più la vostra, colleghi) possa essere non la semplice febbre, ma la febbre perniciosa della ragione della nostra democrazia.

l'ordine del giorno G37, che riguarda un tema che non è stato finora toccato: quello del bilancio di genere. Già l'anno scorso, in occasione del mio intervento sempre sul bilancio interno del Senato, avevo anticipato in Aula che, per iniziativa della Commissione pari opportunità del Senato che lei, signora Presidente, presiede, si era deciso di varare un'iniziativa che è stata accolta dal Presidente del Senato, cioè un'occasione formativa interna del Senato, ma aperta anche anche ai funzionari della Camera dei deputati, per approfondire la tematica del bilancio di genere. Quando si parla di bilancio di genere si intende uno strumento efficace per promuovere un'effettiva parità fra uomini e donne, cioè uno strumento di rilettura della spesa pubblica vista con riguardo all'incidenza delle politiche di genere. L'adozione di una lettura dei documenti contabili nell'ottica di genere infatti consente, da un lato, di introdurre strumenti di verifica dei risultati di gestione delle risorse finanziarie e, dall'altro, di agire da stimolo nel processo di realizzazione dell'equità di genere nei processi organizzativi.

Riguardo a questo vorrei ricordare l'importanza dell'argomento e il fatto che il Senato abbia proprio fatto da apripista per la sperimentazione da applicare al bilancio interno dell'istituzione proprio a seguito dell'iniziativa della Commissione. Vorrei altresì ricordare che a seguito della Conferenza mondiale sulle donne di Pechino, ormai del 1995, il bilancio di genere è diventato uno degli strumenti chiave per la realizzazione delle pari opportunità, e il Parlamento europeo, con la risoluzione n. 30 del 2003, invita tutti gli Stati membri a utilizzare tale strumento come elemento funzionale alla realizzazione della parità. In Italia la direttiva ministeriale del 23 maggio 2007, che reca «Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle pubbliche amministrazioni», prevede l'auspicio che «i bilanci di genere diventino pratica consolidata nell'attività di rendicontazione sociale delle amministrazioni»; il bilancio di genere inizia quindi ad assumere sempre più importanza. La legge n. 39 del 2011 di riforma della legge di contabilità nazionale delega il Governo a introdurre in via sperimentale un bilancio di genere, per la valutazione del diverso impatto delle politiche di bilancio su donne e uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito. retribuito. Pertanto, quello dell'equilibrio nell'ambito professionale, è un aspetto su cui il Senato ha sempre avuto una particolare attenzione e si si propone come apripista per la sperimentazione. Proprio considerando l'estremo interesse suscitato dall'iniziativa, si è tenuto molto recentemente un incontro con i senatori Questori, che hanno dato la disponibilità a verificare - con l'ausilio dell'amministrazione e sin da settembre le modalità in base alle quali la struttura del bilancio interno del Senato possa consentire la sperimentazione e poi l'applicazione dei principi del bilancio di genere. Infatti, la recente legge 7 aprile 2011, n. 39 ha delegato il Governo a introdurre in via sperimentale un bilancio di genere per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini in termini, così come ho detto prima, di denaro, servizi Sarebbe quindi auspicabile che il Consiglio di Presidenza del Senato promuovesse quanto prima, come chiediamo nell'ordine del giorno G37, un impegno da parte del Senato

diretta a verificare le modalità in base alle quali la struttura del bilancio interno del Senato possa consentire l'applicazione dei principi del bilancio di genere, in modo da procedere magari ad una sperimentazione già nel corso dell'esercizio finanziario 2011-2012. Questo rappresenta infatti un piccolo passo per la valutazione dell'impatto, sulle dipendenti e sui dipendenti del Senato, dei principi delle pari opportunità. Ma si tratta di un'iniziativa che potrebbe essere finalizzata a raggiungere un obiettivo più grande, cioè trasmettere all'esterno un messaggio forte di salvaguardia anche nella nostra società e dei valori che la caratterizzano, dell'importanza per il mondo femminile, per le donne (comprese quelle che lavorano nel Senato, che dimostrano grande capacità e professionalità), di giocare un ruolo da protagoniste, per far fronte a sfide come la globalizzazione o l'invecchiamento della popolazione. Per questo è necessario uno sforzo comune con il coinvolgimento di tutti i cittadini, lo abbiamo detto tante volte, giovani e meno giovani, uomini e Proprio le donne possono rappresentare la chiave di volta per dare slancio e dinamismo all'economia, garantendo la coesione sociale di cui la nostra società ha bisogno. Voglio ricordare che abbiamo svolto un grande lavoro come Commissione pari opportunità in vari termini e per molte iniziative, come per esempio la verifica dell'equilibrio nella composizione delle commissioni di esame per i concorsi, la formazione del personale o l'attenzione a un tema importante come quello che viene definito «costi di non parità». Abbiamo discusso in quest'Aula con successo una legge importante, che prevede una norma a garanzia della presenza delle donne nei consigli di amministrazione delle società quotate e delle società pubbliche, una legge che è stata approvata proprio grazie al grande lavoro fatto qui nel Senato e con la collaborazione di tutti. Insomma, cogliamo anche l'opportunità di questo dibattito per affermare che il tema della giusta valorizzazione del mondo femminile è sempre più all'attenzione dei soggetti istituzionali e assume un particolare rilievo sia sia nell'ottica di sviluppare una maggiore attenzione sulle questioni di genere sia nella prospettiva di offrire strumenti concreti per la crescita di specifiche competenze professionali nell'ambito dell'Amministrazione.

l'equilibrio tra la necessità di salvaguardare l'efficienza e l'efficacia del Senato, a garanzia dell'autonomia costituzionale della nostra Assemblea, e la necessità di un un risanamento dei conti che è certamente un'opera poderosa, se pensiamo che il nostro bilancio ha avuto un'evoluzione negli ultimi dieci anni - è stato ricordato anche da tanti altri colleghi - dai quasi 460 milioni ai 602 milioni di quest'anno. Però, questo nostro rispetto non può trasformarsi - lo dico con molta franchezza - in un consenso, in un assenso, in un'accettazione acritica,

lo consideriamo ben poca cosa rispetto a quelle che erano le attese. In ciò non ci aiuta - lo dico con molta franchezza - neppure la tempistica che è stata scelta per esaminare il bilancio del Senato, ossia il fatto che ad agosto, alla vigilia della chiusura dei lavori del Senato, che riprenderanno a metà settembre, si porti un progetto di bilancio (il documento si chiama «Progetto di bilancio») per dare all'Assemblea la possibilità di dare contributi per gli obiettivi che congiuntamente ci stiamo ponendo. ci stiamo ponendo. Non è una gentile concessione quella che si chiede, cioè che il bilancio venga esaminato nei tempi giusti, perché il regolamento interno per l'esame del bilancio del Senato al riguardo parla chiaro: l'articolo 3 prevede che, entro il 28 febbraio, il Consiglio di Presidenza approva il progetto di bilancio e dà mandato ai Questori perché possano raccogliere i documenti e riferire in Assemblea. Tale disposizione non è casuale, perché se si vuole procedere a un giusto risanamento e ad un giusto controllo e trasparenza dei conti della nostra Assemblea, non c'è bisogno del piano industriale (ho sentito parlare del piano industriale in alcuni ordini del giorno): il regolamento già prevede la possibilità di piani di settore che consentono con trasparenza l'organizzazione degli Uffici gestionali per la migliore attività. Sempre il regolamento prevede anche un altro aspetto, perché alla demagogia si sta rispondendo con la demagogia. Sto leggendo in questi giorni sulla stampa qualcosa che

siccome il Senato è più piccolo della Camera, c'è un giornale che ha titolato: «Renato batte Gianfranco». Ora, qualcuno dei senatori Questori vuole gentilmente spiegare a quest'Assemblea che

Il bilancio pluriennale previsionale non è oggetto di deliberazione di quest'Assemblea. Ciò chiarito, possiamo incominciare a parlare di cose serie. Siccome io, più che alle previsioni e agli assestamenti previsionali, credo ai rendiconti e quindi ai conti consuntivi, ricordo che il rendiconto 2010, nell'esame dell'andamento della spesa complessiva, ha stabilito in maniera molto chiara che, tra il 2008 e il 2009 (i due anni in cui è scoppiata la crisi nel nostro Paese di riflesso a una crisi internazionale drammatica), la spesa complessiva del Senato è aumentata dell'1,80 Tra il 2009 e il 2010, altri anni in cui è continuata la crisi, la spesa complessiva è aumentata soltanto dello 0,60 Se poi andiamo ad esaminare questa spesa per aggregati funzionali e togliamo la spesa non comprimibile per il ruolo, che comprende gli emolumenti dei senatori e gli stipendi del personale, la spesa per attività funzionale del Senato tra il 2008 e il 2009 - ci riferiamo sempre ai due anni della crisi economica che sta travagliando il Paese

delle indennità dei parlamentari, la riduzione delle competenze accessorie dei parlamentari e la riduzione degli stipendi più elevati del 5 e del 10 per cento. Poi cosa resta? Resta una rinuncia che è il mancato adeguamento contrattuale. Io ho difficoltà a pensare che in un bilancio di cassa su base annuale una rinuncia rappresenti un risparmio effettivo. Poi abbiamo invece altre voci che si tagliano da un lato e si compensano dall'altro. Abbiamo, per esempio, un risparmio di 300.000 euro per la dematerializzazione degli atti parlamentari e poi, invece, vediamo aumentare il capitolo della stampa degli atti parlamentari da 5.700.000 a 5.950.000 Prevediamo un risparmio di 700.000 euro per la dismissione di alcuni contratti di locazione e poi vediamo aumentare il capitolo dei contratti di locazione da 4.680.000 a 4.782.000 euro.

non solo all'Assemblea, ma anche al resto del Paese, l'impressione che si stia operando con sollecitudine su una razionalizzazione dei costi del Senato.

Alcuni di questi ordini del giorno ce li avete accolti, ma poi sono stati sistematicamente disattesi. Probabilmente qualcuno ha pensato che l'ordine del giorno vale soltanto un giorno...

fummo accolti da sorrisini, ironie, derisioni e denigrazioni. Ora, ci fa piacere vedere che altri autorevoli esponenti e, tra l'altro, grandi esperti economisti stiano venendo sulle nostre posizioni,

delle indennità parlamentari e costituisce una megacommissione, presieduta dal presidente dell'ISTAT e composta da quattro esperti di chiara fama internazionale.

di una riforma della disciplina degli assegni vitalizi; anche loro si sono posti il problema. Allora, bisogna capire qual è la differenza

Francamente è difficile far credere ai Comuni ed alle Regioni - che abbiamo sottoposto a tagli di molti miliardi di euro - che se si prevede l'aumento di una spesa, alla quale poi si rinuncia, quello sia di per sé un risparmio effettivo.

una riforma a costo zero? Miglioriamo la comunicazione intra-istituzionale, perché la dissolvenza della vigilanza e del controllo che i componenti del Senato possono avere sul bilancio interno non aiuta, non agevola.

ai sensi dell'articolo 37 del regolamento interno del Senato, che impone la trasparenza degli atti e delle decisioni prese dal Consiglio di Presidenza, di avere l'elenco degli appalti e degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 100.000 euro,

Se non diamo a questo Palazzo e a questo bilancio trasparenza e comunicazione, non prendetevela con gli italiani e con la zia Iolanda del senatore Ferrara se non ci capiscono.

dell'approssimazione e della mistificazione. Proprio oggi un giornale titola a tutta pagina «La casta impazzita si raddoppia lo stipendio». Questo è un titolo falso, gaglioffo e potenzialmente criminogeno con il quale noi facciamo i conti. Rinvio all'intervento il fatto che i politici italiani non guadagnano più dei colleghi francesi, tedeschi o statunitensi. Ma, come insegnava Goebbels, una menzogna ripetuta 100 volte, 1.000 volte, 1 milione di volte diventa una verità. Allora è più facile credere a certe panzane che circolano in rete, dagli stipendi di 30.000 euro e più, alle auto blu, agli aerei di Stato per ogni singolo parlamentare o benefici (credo mai esistiti, o da tempo aboliti) qualche abile ipocrita si arricchisce a spese della credulità popolare. Tuttavia, attenzione a chiudersi in una sorta di difesa a riccio che, probabilmente, nessuno fuori di qui perché in realtà i cittadini pensano male non perché qualche giornalista cinico e baro racconta quattro balle. Quella è la conseguenza, non la causa. Chiediamoci invece quali sono le cause per cui poi qualche giornalista trova comodo cavalcare la tigre degli umori popolari. Qualche ragione forse c'è. Una prima: i Paesi che citava il senatore Malan sono la prima, la terza e la quinta economia del mondo: noi siamo la dodicesima, con tendenza al ribasso, e tutti gli analisti, senza distinzione di parti politiche, convengono che nel nostro tracollo, nella lentissima ripresa del PIL, nella competitività che scivola oltre il cinquantesimo posto della classifica internazionale, in tutte queste cose il peso della cattiva politica, di ogni colore e di ogni parte, della cattiva amministrazione, è il vero punto debole. Altro aspetto. Il confronto non è non è solo con i nostri colleghi francesi che guadagnano di più, ma anche con il tenore di vita e i consumi della maggior parte dei cittadini italiani onesti, che pagano le tasse e che con quelle tasse pagano anche il nostro stipendio, che faticano più di noi e guadagnano meno di noi, e non certo per loro colpa. Questi non ci perdonano nulla, mentre a generazioni politiche passate sono state perdonate ben altre cose, sull'onda della crescita e, avrebbe detto De Andrè, «lungo un facile vento di sazietà». Se poi aggiungiamo che c'è una questione morale che squassa la classe politica, magari anche perché qualcuno fuori di questa Aula e fuori delle istituzioni, tutte, regola gran parte della spesa pubblica, di 800 miliardi, determinando sacche di malversazione e di spreco, il quadro è completo. Tutto ciò premesso, e consapevoli che, come diceva il senatore Baldassarri, il bilancio del Senato fa 600 milioni su 800 miliardi di spesa pubblica, quindi lo 0,7 per mille del bilancio dello Stato, consapevoli che lo stipendio di tutti noi senatori, tutti insieme, costa ad ogni italiano meno di un euro l'anno; consapevoli di tutto questo, tuttavia chiediamo se si può fare qualcosa di più di quello 0,34 per cento di riduzione, di cui i colleghi senatori Questori si sono anche vantati perché è la prima volta che compare un segno negativo. Sono state dette molte cose:

delle diarie e dei rimborsi, perché stabilite così forfetariamente in effetti diventano un incentivo a non lavorare. Se una persona lavora, è presente, ha gli assistenti, ha gli uffici, spende quei soldi, se li mette in tasca, e questo non va bene. Media europea - perché no - anche per il numero e la retribuzione del personale dipendente. Ho fatto un piccolo conto e ha notato che per ogni senatore il costo del personale dipendente è di 590.000 euro. Mi sembra tanto; forse ce ne sono un po' troppi. La senatrice Leddi aveva evidenziato alcuni possibili sprechi. E anche per la retribuzione individuale trovo sconcertante che lo stesso datore di lavoro ritenga di retribuire di più un incarico meramente d'ordine, meramente esecutivo presso le Camere della Repubblica, piuttosto che per esempio il mestiere di un professore ordinario nell'università di Stato. Si può rivedere il capitolo pensioni, che vale il 30 per cento del bilancio, com'è stato detto. si possono e si devono eliminare tutti i benefici agli ex senatori e si devono limitare i trasporti gratuiti ai soli spostamenti legati al mandato, quindi da e verso Roma, e comunque in modo comprovato legati al mandato. Si possono e si devono contenere e rendere trasparenti i trasferimenti ai Gruppi parlamentari e si devono rendere trasparenti tutti gli acquisti dall'esterno. Diceva il senatore Mascitelli che non gli è stato risposto ad una sua precisa interrogazione; ma queste cose potrebbero essere sul sito. Parliamo di comunicazione istituzionale, e questa lo è: mettiamo sul sito queste informazioni, così le possono vedere tutti. Questa è la trasparenza vera. Un'altra questione riguarda (e arriviamo all'ordine del giorno G13, a firma Musso e D'Alia, che illustro brevemente) la riduzione della produzione e riproduzione cartacea, che oggi è resa inutile dall'uso delle tecnologie info-telematiche. indietro della carta, quando invece possiamo fare le stesse attività, almeno per la gran parte, con il *computer*. Naturalmente molte di queste cose richiedono una volontà politica che probabilmente eccede le possibilità anche del Collegio dei senatori Questori. Per questo, l'ordine del giorno G14, che pure adesso illustro brevemente, sempre a firma Musso e D'Alia, propone di determinare prima il taglio alla dotazione annuale nella misura del 5 per cento, e di conseguenza il saldo del bilancio, e dopo le riduzioni mirate - peraltro non orizzontali, non lineari - su alcune voci di costo. Se il bilancio quest'anno riduce i suoi costi dello «zero virgola», in realtà negli ultimi dieci anni li ha aumentati del 30 contro un aumento del 21 per cento dell'indice dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati: quegli operai e quegli impiegati che ci dicono non soltanto che costiamo troppo, ma soprattutto che, rispetto a quello che costiamo, produciamo molto poco e non diamo l'utilità attesa per il Paese.

in agosto l'attacco all'Italia e all'euro continuerà; la credibilità della politica è un problema, e dentro queste coordinate noi discutiamo il bilancio del Senato. Siamo tutti sotto esame, seriamente. Noi siamo qui in rappresentanza del popolo italiano e per nessun'altra ragione che non sia il bene comune e la dignità delle istituzioni democratiche. si è decisa in quest'Aula - lo ricordo anch'io - una manovra finanziaria che è a carico di tutti gli italiani, soprattutto dei più deboli. Il bilancio del Senato non può non esserne parte. Questa non è una discussione contabile, astratta: è politica. Il bilancio del Senato dipende interamente da noi, è nella piena autonomia dell'Assemblea, non vi sono vincoli di Governo, né di maggioranza, né di approvazione unanime da parte del Consiglio di Presidenza, a mio parere (considero la proposta avanzata nulla più di una istruttoria sullo stato delle cose), né vi sono vincoli di correlazione con quanto ha fatto l'altra Camera. La proposta presentata non è la risposta adeguata alla domanda di rigore e di cambiamento che viene dalla coscienza collettiva e dalla nostra stessa coscienza. È una domanda di sobrietà rivolta alla politica, ai suoi costi e ai suoi comportamenti, la stessa domanda che sta segnando del resto un cambio d'epoca nella vita del mondo, nei valori, nei costumi. Verità, sobrietà, trasparenza, eticità ed essenzialità sono parole che si dicono con facilità, si praticano con difficoltà. Ma è questo che si chiede per ridefinire lo sviluppo, per dare valore alla politica, valore che è essenziale per il destino della democrazia, riscattandolo dalle insidie dell'antipolitica. Signora Presidente, colleghi, questo è il contesto, questa l'urgenza. Il risparmio contenuto nel bilancio 2011 è dello 0,34 per cento: del tutto insufficiente e inaccettabile, e l'andamento previsto nel prossimo triennio conferma semplicemente che le cose non possono continuare così come sono ora. No: saremmo fuori dalla storia di oggi del nostro Paese. Se la crisi economica e finanziaria impone sacrifici a tutti, i primi, non gli ultimi, ad essere chiamati in causa sono i rappresentanti del popolo. Glielo impone il loro ruolo. Come non sentire lo scarto in questo bilancio tra la logica che lo regola e la logica che regola la vita fuori di qui, tra la condizione di vita di milioni di italiani e la nostra condizione di vita, sia pure in modo temporaneo, a tempo, in questa istituzione? La vita delle istituzioni non è separabile dalla vita del Paese. Lo capirono bene i costituenti quando facevano la Costituzione, lo vivevano. Oggi, non diversamente da allora, pur essendo i tempi molto cambiati, una stagione costituente è aperta nell'anima della società italiana, sui fondamenti del suo rapporto con la politica e le istituzioni. In secondo luogo, è urgente riformare, ristrutturare l'intera organizzazione delle istituzioni rappresentative. È tempo di ripensare radicalmente all'organizzazione del Senato e ai suoi servizi, smantellando il reticolo di burocratizzazione, opacità e interessi interni ed esterni che rendono questa organizzazione sempre più pesante e costosa, e non di rado inefficiente. È urgente una drastica riduzione dei costi. Dunque, sobrietà ed essenzialità si impongono. Via i servizi non essenziali, dagli uffici ai ristoranti, dagli affitti a vario titolo ai mezzi di trasporto, dalle spese di rappresentanza alle consulenze. Si abbassino le indennità dei senatori; si aboliscano i vitalizi e le indennità di carica; si ridimensionino i compensi del personale, a partire dalle posizioni apicali, e i finanziamenti ai Gruppi; si elimini ogni spreco; si tolga ogni privilegio. Si tratta di denaro pubblico che appartiene agli italiani. La democrazia costa, certo, ma deve costare nella misura che richiede la democrazia stessa, in coerenza con i suoi valori. Se il tempo tende a consolidare le reciproche convenienze e complicità attorno all'esercizio del potere, la democrazia è appunto il luogo del controllo, dell'affermazione dei principi di giustizia, di uguaglianza, di libertà, del diritto in luogo dei favori. È nelle istituzioni democratiche che devono trasparire innanzitutto i valori essenziali della Repubblica, nell'esercizio delle responsabilità istituzionali e quindi, in questo caso, legislative e nell'organizzazione chiamata a servirle. In terzo luogo - e forse è quello che dà maggiore sofferenza - il tempo è scaduto. Occorre agire ora, senza rinvii. Nessuna continuità oggi può essere ratificata. La nostra responsabilità ci dice che il tempo è adesso. In questi giorni, ancora una volta, il Presidente della Repubblica, riducendo indennità e spese, ha dato l'indirizzo. qualcosa, in questi anni, si è fatto, ma non abbastanza. In altri Parlamenti del mondo - non faccio le comparazioni con gli altri Paesi europei dove si rischia la vita per la democrazia, ogni parola, ogni decisione si paga a caro prezzo. Qual è il prezzo che noi siamo chiamati a pagare, se non quello della coerenza e della responsabilità? Guai a non capire che cosa è in gioco oggi in Italia e nelle Aule parlamentari. Questo bilancio è lo specchio di ciò che siamo, ma noi abbiamo bisogno di decidere da qui in avanti quale sarà lo specchio di ciò che vogliamo essere e di come in tutti i settori potrebbe essere l'Italia. Occorre cioè una forte iniziativa politica che ristrutturi la politica, e possiamo cominciare dalla ristrutturazione del Senato. In queste ore, il Senato e la Camera degli Stati Uniti, il Congresso affrontano questioni decisive per il mondo intero, noi semplicemente il bilancio del Senato della Repubblica, ma gli interrogativi sono gli stessi. La crisi è gravissima; chi la pagherà, tra i ricchi ed i poveri? Occorre il coraggio del rigore, a partire da noi stessi e la politica sarà credibile solo se noi saremo credibili. Dobbiamo dunque cominciare da noi, dobbiamo essere esigenti innanzitutto con noi stessi; davvero nessuno, nessun altro può farlo al nostro posto, ora. Colleghi senatori, perdonate, ma a me sembra così elementare.

giorni fa, nell'approvare il bilancio interno che oggi l'Aula esamina e che voteremo domani mattina, ha previsto una serie di tagli alle spese, sulla strada del contenimento dei costi che contraddistingue nel corso di questa legislatura

gli effetti che sono stati prodotti dalla Presidenza dell'attuale presidente Schifani - riuscendo ad invertire una tendenza, quel *trend* di crescita del fabbisogno che era inesorabilmente in crescita fino al 2008. Le riduzioni previste riguardano - vorrei ricordarlo perché altrimenti ci perdiamo in tante discussioni che riguardano questo come altri mondi

e solo grazie ed in virtù di un accordo ampio, di condivisione e di rappresentanza sindacale tra i dipendenti del Senato e la nostra Presidenza, con la presidente Mauro delegata a questo scopo, siamo riusciti ad incidere su una delle spese più rigide e più inamovibili del bilancio, cioè quella del personale.

voce rilevante per quei risparmi che andiamo a strutturare, e neanche così lentamente, nella progressione e nella proiezione dei bilanci futuri. Analogamente lo stesso contributo viene applicato ai vitalizi degli ex senatori che si trovano nelle medesime condizioni, che sono assai pochi per la verità. verità. I dati e le cifre che ci ha illustrato così bene ieri il senatore Malan hanno messo in evidenza e ricordato a tutti noi alcune verità che molti hanno invece interesse a far dimenticare, spesso all'interno di interventi anche aulici e ispirati che, però, non tengono conto della realtà e della verità e offrono una verità distorta. Per effetto delle decisioni dei mesi scorsi e grazie all'approvazione di questo bilancio, il Senato vedrà ridotti i suoi costi complessivamente - e lo ricordo in particolare al senatore Giaretta - di 120 milioni di euro per il triennio 2011-2014. triennio 2011-2014. Ha ragione il senatore Morando quando richiama alla programmazione e alla pluriennalità del nostro bilancio, e ciò è stato ricordato benissimo anche dal senatore Mascitelli, ma il dato è certamente questo: gli atti e le decisioni del Consiglio di Presidenza, così come nei mesi scorsi con il recepimento della manovra economica, hanno comunque già determinato questo tipo di risparmio. Nel momento in cui il Paese vive davvero la sua più dura crisi economica, e su questo hanno ragione tutti i senatori che lo hanno ricordato, ha certamente un valore rilevante collegare strettamente l'attività e il ruolo che qua dentro svolgiamo alla situazione che vive il Paese. Non c'è un Senato o un Parlamento distante o distaccato dalla vita del Paese: chi lo dice e chi lo evoca chi lo dice e chi lo evoca è perché ha interesse ad indebolire sempre più questo Senato e questo Parlamento nella sua azione di controllo, di possibile controllo sull'intera attività normativa proposta dal Governo. E oltre il *continuum* costituzionalmente garantito ai Governi e alle loro maggioranze, oggi abbiamo la necessità di recuperare quel *continuum*, già costituzionalmente garantito proprio dalle guarentigie dei parlamentari, tra rappresentati e rappresentanti. E noi ci dimentichiamo sempre di questo dettaglio, perché invochiamo una nuova Costituente, ogni volta abbiamo qualcosa da ricostituire o da riformare, e ci dimentichiamo che chi ha lavorato prima di noi, provenendo da esperienze, quelle sì, drammatiche, come quando il Paese usciva dalla guerra e dal fascismo, ha fortemente voluto garantire al ruolo del rappresentante dei cittadini quelle prerogative che voi, un pezzo alla volta, una picconata al giorno, avete oramai irrimediabilmente distrutto, al punto che al punto che potete oggi dire (è vero, convintamente, e forse anche con qualche ragione) che questo Parlamento è totalmente scollegato dal resto del Paese. Una cosa è sicura: che quel resto del Paese non lo rappresentate voi, perché voi rappresentereste quel Paese nel momento in cui, oltre che a preoccuparvi di come tenere la barra dritta sulla prospettiva della tenuta dei conti e della crescita economica, riusciste a dotare questo Paese, che voi ed noi amiamo, di uno strumento parlamentare forte, vero, che sappia fare il proprio lavoro e sia nelle condizioni di farlo. Ma a voi questo forse non interessa, mentre invece dovremmo molto preoccuparci di questo. Ma sono sicura non è questo il caso in cui noi dobbiamo dividerci. Non c'è un noi e un voi in questa situazione: c'è un "tutti noi", che dobbiamo difendere il valore di questa democrazia e questa democrazia la si difende raccogliendo la sfida che ha lanciato il Presidente della Repubblica. Do merito al Presidente della Repubblica di aver lanciato un'importantissima sfida: lui ha rinunciato a circa 100 euro di aumento del suo stipendio; ma noi abbiamo capito che nonostante questo risparmio così piccolo, dietro c'era un appello importante, che noi abbiamo raccolto, per difendere questa democrazia contenendone i costi. Questo sì: non senza costi, ma contenendone i costi. Difendere questa democrazia risparmiando, perché si potrà ancora risparmiare, ne sono certa e i nostri senatori Questori, che hanno già svolto un importantissimo lavoro, continueranno a svolgerlo. Il Consiglio di Presidenza, che si sente rappresentante di tutti i senatori e a sua volta quindi di tutti cittadini, ha la responsabilità di sostenere gli sforzi che la Presidenza di questo Senato, il Presidente e i Vice Presidenti stanno compiendo per rendere tutto questo possibile, concreto, tangibile. Siamo sicuri che ancora tanto si può e si potrà fare, e lo faremo, perché tra tra le chiacchiere, anche ispirate, e la realtà, la differenza sta tra chi fa e chi non fa; e questo Senato, quest'Aula, tutti noi, in questa legislatura qualcosa abbiamo e quel *trend* che ricordavo all'inizio del mio intervento è stato bloccato, invertito. Questo è quello che vorrei ricordare al senatore Molinari, che ieri si prodigava in un attacco alla cerimonia del Ventaglio. Vede, se è vero, come è vero, signora Presidente, che nel bilancio del Senato la voce senatori e tutte le competenze ad essi riferite - che vi prego di considerate al netto, senza cadere anche noi nell'errore voluto e in malafede di chi paragona il nostro stipendio lordo con gli stipendi netti dei parlamentari degli altri Paesi

del blocco del *turnover* che non aveva precedenti (così come non aveva precedenti, prima del 2008, il passaggio al regime contributivo per i dipendenti del Senato, che invece fino al giorno prima godevano del regime retributivo: e questo non l'avevamo fatto noi). Quindi, le spese su cui dobbiamo certo ancora lavorare sono quelle di funzionamento del Senato. Su questo ha perfettamente ragione chi lo ha ricordato prima di me. Faremmo bene, per esempio, vista la richiesta così forte che il senatore Mascitelli ci ha ancora ricordato nel suo intervento, ad avvalerci degli strumenti moderni che la pubblica amministrazione, per esempio, è riuscita a trovare nel suo sforzo di contenimento dei costi affidando a CONSIP il ruolo di assistenza tecnica per svolgere e aiutarci a svolgere le gare entro parametri di mercato, già contrattati dalla pubblica amministrazione e per la pubblica amministrazione. Concludo quindi ricordando al senatore Molinari che non sono favorevole ad abolire la borbonica cerimonia del Ventaglio, che peraltro quest'anno per la prima volta non è costata un euro, non è costata un euro, perché il presidente Schifani ha preteso di farla semplicemente nella sala Zuccari, senza nessun tipo di costo e senza offrire neanche un bicchiere d'acqua ai giornalisti che intervenivano a quella cerimonia; non sono per abbandonare una cerimonia che ricorda la tradizione e la condivisione con la stampa, quella sì, molto competente e seria, che tutti vorremmo avere in questo Paese. avere in questo Paese. Al senatore Molinari ricordo semplicemente che la differenza tra le cose che lui dice e la realtà è che il Presidente del Senato, Renato Schifani, tutte queste cose, tutti questi tagli li ha fatti. Vedremo se sarà capace di farli anche lui.

tra il 31 luglio ed oggi, alcune decine di migliaia di lavoratori escono dalla cassa integrazione e probabilmente, per errori fatti dal nostro Ministro dell'economia, non riceveranno la pensione per i prepensionamenti, perché ne erano previsti 10.000 e forse sono di più, molti di più.

Io penso che noi facciamo bene a ridurre fortemente i costi della politica, ma se a questi lavoratori, come quello che oggi ha tentato di suicidarsi di suicidarsi a Napoli, non diamo risposta, noi non saremo capiti, perché il nostro mestiere è anche risolvere le questioni di cassa integrazione, di prepensionamenti, di disagio.

non è bello. Noi ci occupiamo di tante cose; sarebbe bene che questo Parlamento si occupasse con un po' più di precisione delle condizioni di queste persone, che - quelle sì - ci chiedono che cosa facciamo

Lei ha quindi fatto una serie di valutazioni e di commenti politici, che spettano al ruolo del parlamentare.